1 marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha nominato il professor Roberto CINGOLANI Ministro della transizione ecologica, il professor Enrico GIOVANNINI Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'onorevole Dario FRANCESCHINI Ministro della cultura e l'onorevole Massimo GARAVAGLIA Ministro del turismo.

il provvedimento in esame reca ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione della Covid-19, nonché disposizioni in merito allo svolgimento di elezioni per l'anno 2021. Il decreto-legge si compone di sei articoli. L'articolo 1, ai commi 1 e 2, differisce dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 il termine per l'applicabilità delle misure restrittive contenute all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020,

esame, in seguito all'approvazione di tale emendamento, prevede fino al 27 marzo 2021 il divieto, già in vigore, di ogni spostamento tra Regioni e Province autonome diverse, con l'eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Inoltre, fino a tale data, è consentito in ambito in ambito comunale nella zona arancione lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa. 4-*ter*. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.»; Infine, si prevede l'inserimento nell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 delle denominazioni «zona gialla», «zona arancione», «zona rossa» e «zona bianca», già utilizzate nei provvedimenti attuativi per definire le zone caratterizzate da diverse tipologie di scenario (1, 2 e 3), differente grado di rischio epidemiologico e con una determinata incidenza settimanale dei contagi ogni 100.000 abitanti, secondo i parametri già disciplinati ai commi 16-*quater* e 16-*quinquies* del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 33. L'articolo 2 prevede che la violazione delle disposizioni dell'articolo 1 sia sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione ha approvato un emendamento volto a specificare che, in linea con quanto previsto con il decreto-legge n. 33 del 2020, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari ufficiali e agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle Regioni, alle Province e ai Comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari ufficiali e da agenti rispettivamente delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Inoltre, con l'approvazione di due identici emendamenti, si stabilisce che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica per la Covid-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi culturali e sociali, adottati nell'ambito della misura di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo e analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento anche occasionale o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie di predetti enti. L'articolo 3 concerne alcuni profili dell'attività di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2. In particolare, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, è istituita una piattaforma informativa nazionale per agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione e relativo tracciamento. La piattaforma è predisposta e gestita dal Commissario straordinario per l'attuazione del coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il quale, avvalendosi prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica, opera in modo coordinato con i diversi soggetti istituzionali coinvolti e, d'intesa con il Ministero della salute e il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sullo stato di attuazione del piano strategico. Le diverse fasi della vaccinazione sono affidate alle Regioni e alle Province autonome che si avvalgono dei propri sistemi informativi e vaccinali in qualità di titolari del trattamento. qualora il sistema informativo vaccinale di una Regione o di una Provincia autonoma non risulti adeguato, su istanza del medesimo ente, la piattaforma nazionale esegue, in regime di sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse. Le Regioni e Province autonome, attraverso i propri sistemi informativi o attraverso la piattaforma nazionale, trasmettono al Ministero della salute tutte le informazioni relative alla somministrazione dei vaccini sulla base individuale, in conformità del decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2018, istitutivo dell'Anagrafe nazionale dei vaccini. Sono tenute inoltre a trasmettere i dati relativi alle prenotazioni delle vaccinazioni in forma aggregata al Ministero della salute il quale renderà disponibili alla piattaforma nazionale strumenti di monitoraggio sia delle prenotazioni, sia delle somministrazione dei vaccini. Si prevede inoltre che al fine di consentire lo svolgimento di attività di sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologica, il Ministro della salute trasmette all'Istituto superiore di sanità i dati individuati relativi ai soggetti cui è stata somministrata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale dei vaccini. È infine autorizzata la spesa di 966.000 euro per il 2021 per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e l'applicazione dell'Anagrafe nazionale vaccini. L'articolo 4 dispone in merito allo svolgimento di elezioni per l'anno 2021. Nello specifico si prevede che le elezioni suppletive per seggi della Camera e del Senato dichiarati vacanti entro il 28 febbraio del 2021 si svolgano entro il 20 maggio 2021. A tale fine è novellato l'articolo 31-*quater* del decreto-legge n. 137 decreto ristori, il quale stabiliva, nel testo previgente, che le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato, dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020, si svolgessero entro il 31 marzo 2021. Anche il termine entro il quale dovranno svolgersi le elezioni degli organi elettivi dei Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, già oggetto di prima proroga, operata dall'articolo 1,

Con riguardo a questo articolo, in Commissione è stato approvato un emendamento che estende anche all'anno 2021 l'applicazione della norma di cui all'articolo 1-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 26 del 2020, che aveva stabilito, per le elezioni nelle Regioni a statuto ordinario del 2020, che il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e delle candidature, a causa della pandemia da Covid-19, fosse ridotto a un terzo. Inoltre, tale proposta estende anche al 2021 la possibilità per ciascuna Regione di prevedere disposizioni normative diverse da quelle contenute nel comma 5 del medesimo articolo, per prevenire e ridurre il rischio di contagio da Covid-19. L'articolo 5 novella l'articolo

decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio ha differito lo stato di emergenza al 30 aprile prossimo e così il decreto-legge n. 2 del 2021, che oggi ci apprestiamo a convertire in legge, differisce allo stesso termine l'applicabilità di tutte le misure restrittive, che al momento appaiono ancora necessarie a contenere il rischio di diffusione del contagio da Covid-19. L'intervento normativo del nuovo Governo e le discussioni nelle Commissioni competenti sul decreto-legge in esame, che ricordiamo è in vigore dal 14 gennaio, hanno reso possibili delle piccole modifiche, rendendolo più uniforme e armonioso, riguardo all'indicazione delle date di termine delle misure, e definendo meglio e più semplicemente il contenuto della denominazione delle zone ad alto rischio di contagio, fino a quelle con un livello di rischio moderato e di rischio basso, con l'indicazione chiara dei limiti di spostamento in ambito regionale e comunale. È ampliata la fattispecie del passaggio del territorio regionale dalla zona gialla a quella arancione, prospettando anche una zona bianca, libera da ogni limitazione valevole per le zone rosse, arancioni e gialle, ferma restando l'applicazione di determinate misure e protocolli. Il decreto-legge prevede, all'articolo 2, le sanzioni nel caso di violazione delle misure di contenimento del contagio, delineandone anche il procedimento di applicazione, con un rinvio esplicito all'apparato sanzionatorio vigente. Infatti, a seconda della violazione commessa, si dispongono sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie e, tra queste, mi pare utile ricordare il rinvio alla pena contravvenzionale dell'inosservanza di «un ordine legalmente dato, per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo», *ex* articolo 260 del Testo unico delle leggi sanitarie (nel caso in cui il fatto non integri un delitto colposo contro la salute pubblica o comunque un più grave reato), l'inosservanza della quarantena, e per cui la sanzione consiste nell'arresto da tre a diciotto mesi e nell'ammenda da 500 a 5.000 euro, con l'esclusione, per la combinatoria delle pene congiunte, della possibilità di oblazione. Vengono definiti poi alcuni profili dell'attività vaccinale, con la previsione dell'istituzione di una piattaforma informativa nazionale per agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e di tutti i materiali di supporto alla somministrazione e il tracciamento relativo; il raccordo con l'Anagrafe nazionale dei vaccini, istituita con il decreto ministeriale del 17 settembre 2018; l'informazione da parte del commissario straordinario (che oggi riconosciamo nel generale Figliuolo, a cui vanno i nostri auguri di buon lavoro), d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro degli affari regionali e delle autonomie, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sullo stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini in oggetto. Il decreto-legge poi, all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, posticipa le elezioni suppletive per i seggi dichiarati vacanti di Camera e Senato, che devono svolgersi entro il 20 maggio. Allo stesso modo, entro la stessa data, vengono differite le elezioni per i Comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose, prorogando nelle more la durata della gestione della Commissione straordinaria in deroga alla normativa vigente. Inoltre, all'articolo 5, prevede l'estensione, fino al 30 aprile, della validità dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, nonché l'efficacia dei titoli di soggiorno in materia di immigrazione, ricomprendendo quindi nel regime di proroga quelli in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021. un decreto-legge quindi che continua a prevedere proroghe a quelle misure restrittive, molto stringenti in alcuni casi, adottate fin da subito con un susseguirsi di per far fronte ad una situazione nuova ed improvvisa, che ha colto il mondo di sorpresa; misure che hanno condizionato in questi mesi le libertà personali di ognuno di noi. limitato il diritto di circolare liberamente per strade urbane, parchi, spazi pubblici, il diritto di frequentare luoghi di svago e divertimento, il diritto di usufruire dei servizi educativi e della didattica in presenza da parte dei nostri ragazzi e finanche il diritto di lavorare. Infatti, se la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti hanno risolto temporaneamente la situazione lavorativa di molti dipendenti, è innegabile che in tempi brevi serve un intervento audace sulle politiche attive del lavoro. È innegabile anche la crisi profonda di molte attività di imprese professionali e artigianali, che non hanno superato le gravi difficoltà dovute alla limitazione e alla sospensione delle stesse attività, con gravissimo danno economico, ma in particolar modo danno sociale, dove la stessa dignità delle persone è stata purtroppo sacrificata, senza i dovuti provvedimenti, non di ristoro, ma di apertura e soluzione di tavoli di crisi a vari livelli. Tuttavia, colleghi, non è il tempo delle recriminazioni e quindi è corretto e onesto intellettualmente dire che le misure introdotte con i vari provvedimenti di cosiddetta prevenzione dell'emergenza epidemiologica, malgrado le conseguenze che sono visibili a tutti e per cui, in virtù di una speculazione mediatica di propaganda, abbiamo in questi mesi sentito dire tutto e il contrario di tutto, sono servite a tutelare un diritto fondamentale e assoluto garantito dalla nostra Carta costituzionale: il diritto alla salute di tutti noi. Di fronte a un virus sconosciuto che si è diffuso velocemente in tutto il mondo e così anche nelle nostre Regioni italiane è stato necessario intervenire - e lo è ancora - con limitazioni ad alcuni diritti di libertà, con uno strumento normativo straordinario e che ora con questo decreto proseguono. Vi è però una differenza riguardo a prima e cioè che contemporaneamente stanno cambiando degli equilibri, che sicuramente ci permetteranno di gestire con una visione diversa ogni situazione sanitaria e di agire in modo coordinato per attenuare, di conseguenza, le ripercussioni socio-economiche nelle Regioni del Nord, come nelle Regioni del Sud. Penso ad esempio alla mia Calabria, dove urge una nuova gestione con maggiore competenza del Piano vaccinale, la cui velocizzazione, ma soprattutto la migliore organizzazione anche a livello di interlocuzione e confronto in Europa e con le Regioni, è fondamentale per affrontare meglio nell'immediato, e superare definitivamente poi, questo periodo di pandemia che ha cambiato ormai, forse in modo irrecuperabile, le nostre abitudini di vita. Mi sento di dire però che non potrà mai cambiare la nostra voglia di andare avanti, creando le condizioni di fiducia nel futuro per tutti i nostri giovani, nei cui confronti abbiamo il dovere di garantire la possibilità di affrontare da protagonisti le sfide dei prossimi anni. Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghe e colleghi, l'incidenza dell'epidemia nella quasi totalità delle Regioni italiane è ancora molto preoccupante ed elevata. Ciò evidenzia l'esigenza, soddisfatta dal decreto in esame, di adottare ancora misure rigorose di contrasto e di contenimento alla diffusione dell'epidemia. Il differimento al 31 aprile 2021 del termine dell'adozione di misure straordinarie ai fini del contenimento della diffusione della Covid-19 e della riduzione del rischio di contagio riguardanti limitazioni agli spostamenti ed assembramenti di persone, nonché lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali trova giustificazione nell'attuale evoluzione del quadro epidemiologico nel quale - si osserva - la curva dei contagi resta sempre troppo elevata. Anzi, per la seconda settimana consecutiva si registra un aumento dei contagi del 22 in più rispetto a domenica scorsa. Ciò denota che la continua circolazione del virus è in atto a causa soprattutto delle particolari caratteristiche delle nuove varianti. Pertanto, Pertanto, la gestione di una nuova fase dell'emergenza epidemiologica e, come ricordato, il carattere particolarmente diffuso del virus non possono che richiede ancora l'adozione di urgenti e stringenti misure di intervento.

profonda gratitudine per il lavoro svolto e per le dure e difficili scelte che ha dovuto adottare nel periodo più buio della nostra storia repubblicana. Il sistema dei colori, tanto vituperato in quest'Aula, ha scongiurato un'ipotesi di *lockdown* duro che avrebbe avuto conseguenze ancora più pesanti. Va soprattutto ricordato che siamo uno dei pochi Paesi che è riuscito a evitare questo *lockdown*, a differenza dei tanti altri che vengono sempre citati, come Regno Unito e Germania, che hanno dovuto necessariamente fare ricorso ad un *lockdown* duro, lungo e generalizzato. In virtù dell'elevata diffusione delle nuove varianti, tuttavia, è necessario intervenire per effettuare le dovute correzioni e i consequenziali adeguamenti al nuovo scenario epidemiologico. Prima di analizzare le disposizioni relative al piano vaccinale, vorrei soffermarmi sull'articolo 4 del decreto-legge, che interviene sui termini di svolgimento delle elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e su quelli relativi alle elezioni degli organi elettivi nei Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, nonché sul rinnovo delle elezioni comunali a seguito di eventuale annullamento dei risultati elettorali di alcune sezioni. L'articolo 4 stabilisce che tali elezioni devono svolgersi entro il 20 maggio 2021. Certamente la misura dispone una sospensione della volontà popolare di esercitare il diritto di voto costituzionalmente garantito. Si tratta di una misura pesante che incide sull'interesse primario sancito dalla Costituzione, ovviamente meritevole di tutela, ma che trova giustificazione nell'esigenza del contenimento dei Muovere migliaia di persone per le consultazioni elettorali, come ricordato anche dal Presidente della Repubblica anche nella formazione di questo Governo, potrebbe avere delle conseguenze non accettabili con riferimento alla situazione epidemiologica in atto. Pertanto, la posticipazione delle consultazioni elettorali resta necessaria per la gravità della situazione epidemiologica. Infine, il decreto in esame, all'articolo 3, istituisce una piattaforma informativa nazionale che ha come scopo primario quello di assicurare l'ottimizzazione dell'attività di distribuzione delle dosi vaccinali, dei dispositivi e dei materiali a supporto della somministrazione sul territorio nazionale. Questa piattaforma sarà indispensabile per garantire su tutto il territorio l'uniforme attuazione del piano strategico, ma soprattutto per evitare eventuali discriminazioni di trattamento tra i Comuni e i cittadini italiani. Certo, questo non basta. Anzi, oggi i principali sforzi del nuovo Governo devono essere indirizzati al piano vaccinale, all'urgenza di mettere con immediatezza in atto la fase 2 del programma. Le originarie previsioni del piano strategico della vaccinazione anti SARS-CoV-2 dovranno essere messe in relazione alla effettiva disponibilità di vaccini, a causa della mancata consegna delle dosi. E su questo punto auspico che il presidente Draghi eserciti la dovuta pressione anche sulle istituzioni dell'Unione europea. Non possiamo essere ostaggi di scelte arbitrarie delle case farmaceutiche. La priorità del Paese è quella di garantire subito i vaccini. Inoltre, bisogna tener conto delle limitazioni previste per la somministrazione del vaccino prodotto da AstraZeneca, idoneo soltanto per i soggetti al di sotto dei sessantacinque anni di età, che risultano cioè esclusi dalle prime fasi del piano vaccinale originario. signor Presidente, l'unica cosa da fare è agire in fretta, aumentare le somministrazioni giornaliere sfruttando qualsiasi luogo possibile e idoneo per accelerare la campagna vaccinale. L'unica arma che abbiamo a disposizione per sconfiggere questo terribile virus è il vaccino e immunizzare in fretta ampie fasce di popolazione significa incidere sulla sua circolazione *(Applausi)*. Signor Presidente, colleghi, ieri abbiamo potuto leggere il primo DPCM dell'era Draghi. Non vi nascondo che ero un po' incuriosito di vedere cosa avrebbe potuto produrre il Governo dei migliori. Ebbene, leggendolo abbiamo potuto vedere che in sostanza non è cambiato nulla: il vecchio articolo 12 adesso è l'articolo 3; il vecchio articolo 5 è diviso a metà tra il nuovo articolo 5 e il nuovo articolo 6; il vecchio lunghissimo articolo 1 è diluito nei più snelli articoli 1, 2, 7, 9, 10 e 11. Tuttavia, colleghi, ci sono scritte esattamente le stesse cose. L'ultimo DPCM di Conte del 14 gennaio e il nuovo DPCM del Governo dei migliori si somigliano in tutto e per tutto: stessi colori, stesse parole, stessi contenuti e purtroppo stessa filosofia che si potrebbe riassumere in tre semplici chiudere tutto, chiudere tutto, chiudere tutto! Questa è la nuova filosofia, esattamente identica a quella precedente al Governo dei migliori.

che l'articolo 13 della Costituzione afferma sempre che la libertà personale è inviolabile; che l'articolo 16 della Costituzione stabilisce che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salve le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza; che l'articolo 17 afferma sempre che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente; che l'articolo 34 stabilisce sempre che la scuola è aperta a tutti; che l'articolo 30 dice sempre che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni

Eppure, cari colleghi, molti di voi, soprattutto coloro che oggi fanno parte della minoranza della maggioranza,

strumento discutibile, di usurpazione dei poteri, di scandalo incostituzionale, di Costituzione calpestata limitazione delle libertà coi DPCM che esautorano il Parlamento. Queste sono soltanto alcune delle citazioni di coloro che prima gridavano allo scandalo e oggi si sono completamente silenziati, accettando quindi questi strumenti che rappresentano - a nostro giudizio il nuovo che avanza, ma semplicemente una continuità assoluta con il vecchio Governo Conte II, che potremmo tranquillamente chiamare, anziché Governo Draghi, Governo Conte-*ter.* Non devo ricordare a voi gli allarmi lanciati da autorevoli costituzionalisti come Sabino Cassese, che ha dichiarato recentemente che prima o poi anche la Consulta boccerà le misure anti-Covid e ha messo in rilievo che con questi DPCM si invade un campo riservato all'azione legislativa, tra l'altro in modo parossistico, creando confusione tra i cittadini. E non vi devo ricordare nemmeno la recente pronuncia del tribunale di Roma del 16 dicembre dell'anno scorso, la quale ha stabilito che il DPCM il DPCM è un atto amministrativo che non può restringere le libertà fondamentali, nemmeno - si badi bene - se a legittimarlo è un atto che ha forma di legge. Di tutto questo, il nuovo DPCM del Governo, che abbiamo potuto leggere ieri, ha fatto semplicemente carta straccia. Cari colleghi, noi non siamo contrari che si adottino misure per contenere la calamità che ha colpito l'Italia e il mondo intero - ci mancherebbe altro ma riteniamo che queste misure che incidono sulle libertà fondamentali sancite dalla nostra Costituzione debbano essere discusse nella sede opportuna e appropriata, che è il Parlamento. E mi riferisco anche all'alto richiamo del Presidente del Senato di poche settimane fa: questa è la sede in cui si devono discutere misure che incidono sulla libertà personale, sulla libertà di movimento, sulla libertà di iniziativa economica, sulla libertà di poter vivere una vita degna di questo nome. si deve decidere soprattutto in modo ragionevole come si può intervenire su quella che non è più un'emergenza come poteva esserlo un anno fa, perché emergenza vuol dire una circostanza imprevista e imprevedibile. La seconda ondata non solo non era imprevista né imprevedibile, ma era addirittura annunciata. Eppure, il Governo precedente,

in una situazione che è a tutti nota ed era prevista. Dobbiamo immaginare che non si può chiudere sempre e soltanto tutto, tra l'altro colpevolizzando soltanto alcune determinate categorie. Non ha senso continuare a sostenere che i ristoranti possono rimanere aperti a pranzo, ma devono chiudere la sera: che senso ha? Se il virus circola a pranzo, circola ugualmente anche la sera. Occorre stabilire delle regole, occorrono dei protocolli, come si era anche immaginato di poter fare. Tutte le attività economiche - bar, ristoranti, cinema, teatri, palestre e impianti sportivi

prescrizioni per la tutela della salute devono poter continuare e riprendere la loro attività. Questo è quello che diciamo noi di Fratelli d'Italia. Certo, Certo, vorremmo che le mascherine fossero vere e non farlocche, come quelle che ha comprato l'ex - per fortuna - commissario Arcuri. vorremmo che ci fossero dei controlli sugli acquisti che facciamo per le protezioni che destiniamo ai nostri sanitari e a tutti i cittadini. che ci si interrogasse - ad esempio - sul trasporto pubblico, perché è chiaro che il contagio è lì; ma lì non si interviene. E vorremmo anche che ci si interrogasse sul perché - esponenti di Fratelli d'Italia che in sicurezza fanno una conferenza stampa vengono multati e, nello stesso tempo, assistiamo a spettacoli incredibili di centinaia e centinaia di migranti ammassati, nei confronti dei quali nessuno interviene. È iscritta a parlare la senatrice Pirovano. Ne ha facoltà. Presidente, membri del Governo, devo dire che la sensazione di spaesamento

Mi sembra - secondo una famosa frase di uno dei romanzi più noti d'Italia - che tutto cambi perché in realtà nulla cambi. Questa sensazione è cominciata la settimana scorsa con la fiducia; davanti a una maggioranza così allargata, non si capiva quale necessità ci fosse della fiducia. *(Brusio)*. PRESIDENTE. Posso chiedere ai colleghi che sono vicini alla senatrice Binetti di abbassare il tono della voce, cortesemente?

con tempi così veloci che le Commissioni non hanno avuto il tempo né studiarlo, né di affrontarlo, né di subemendarlo. Ci siamo trovati davanti a un vero e proprio *blitz*. questa operazione fosse stata messa in atto dal Governo precedente, l'avremmo data per acquisita come una delle classiche manovre per cui il Parlamento viene decisamente sottovalutato dal Governo. Ma da questo Governo noi ci aspettiamo qualcosa di più: una delle cose che ci aspettiamo veramente tutti è una maggiore valorizzazione del Parlamento, del ruolo di ognuno di noi, positivo, concreto, incisivo. Questa cosa è mancata nel Conte-*bis* e speravamo tutti potesse farsi realtà nel Governo Draghi. Detto questo, un'altra cosa che mi interessa sottolineare è che in realtà, poi, questo decreto-legge non è altro che una mappa a colori, in cui magari sussiste una maggiore precisione chirurgica nel definire i contorni delle varie zone. Abbiamo visto apparire, tra i tanti colori (il giallo, l'arancione e il rosso), anche l'arancione rafforzato, che pone vincoli, che in qualche modo limita le libertà e rende a noi più difficile capire esattamente cosa si possa o no fare.

il dottor Arcuri sia passato ad altre funzioni e che al controllo e alla predisposizione del piano vaccinale sia stata chiamata una persona che, in linea di principio, dovrebbe avere grande esperienza nell'organizzazione di un sistema ampio.

ma perché la contraddizione continua a essere fortissima anche nella comunicazione che viene data attraverso gli organi di stampa.

proprio per evitare lo stato di confusione. Ma se noi pensiamo che tutto resta uguale nelle modalità con cui si svolgono gli interventi, l'unica speranza è che il vaccino arrivi in tempo reale e a tutti, tenendo conto di di alcune precedenze. Abbiamo sottolineato ieri, in occasione della giornata delle malattie rare, quanto fosse importante che i soggetti con malattie rare venissero considerati tra i soggetti fragili e avessero diritto al vaccino.

Non sappiamo nulla dell'anagrafe vaccinale. Eppure, sappiamo quanto sarà importante, a un certo punto, poter testimoniare e garantire che una persona si è vaccinata, perché ciò determinerà una sorta di patente

nulla. Gli esperti ci danno informazioni difformi e le interrogazioni che abbiamo presentato non hanno avuto risposta; prego l'attuale Governo di assumere come una sfida positiva la necessità di rispondere alle interrogazioni presentate dai parlamentari, perché ogni interrogazione è un problema che coinvolge una parte della popolazione. Noi siamo in attesa

Signor Presidente, membri del Governo, anche ciò rappresenta un elemento di dubbio rispetto al modo con cui l'Europa sta gestendo quest'operazione. Tutti noi siamo europeisti convinti e vogliamo muoverci nella solidarietà complessiva che garantisce la salute di tutti, perché mai come in questo caso è evidente che o ci si salva tutti oppure basta una variante qualunque sfuggita al controllo per rilanciare una nuova ondata di epidemia. Ma la strigliata che il presidente Draghi sembra abbia fatto in Europa nel suo primo atto pubblico come Presidente del Consiglio, proprio proprio in merito ai vaccini, la dice lunga sul fatto che probabilmente la gestione precedente non era stata né così soddisfacente né così capace di garantire tutti i Paesi europei. Questi sono i veri problemi su cui la gente attende risposta. Tutto il resto ormai dipende da questo. Paradossalmente, tutta la situazione anche economica, tutta la situazione scolastica, la vita dei nostri ragazzi, la possibilità per loro di accedere a una formazione intellettuale rigorosa, solida, auspicabile anche nella prospettiva di futuro dipende dal vaccino: vaccino sì o vaccino no. E allora, colleghi, sul tema del vaccino noi vogliamo idee che chiare, ben distinte e soprattutto tradotte in una operatività concreta. Il DPCM nulla ci dice su questo: continua a muovere lo scacchiere della divisione degli spazi, ma non garantisce che davvero alle persone i vaccini arrivino nei momenti opportuni, nelle dosi opportune e con la scadenza opportuna. Anche per questo credo che noi un briciolo di perplessità continuiamo a mantenere anche rispetto a questo Governo.

Nei sei articoli che compongono il provvedimento sono contenuti importanti disposizioni necessarie ad affrontare l'emergenza sanitaria nazionale dovuta al diffondersi del coronavirus. Il decreto-legge in discussione si è reso necessario a causa dell'andamento dei dati sulla situazione sanitaria dovuta alla pandemia, ad inizio gennaio di quest'anno, e in particolare ai numeri riferiti ai soggetti risultati positivi al tampone, all'indice RT di contagio, alla pressione sulle strutture sanitarie (in special modo ai reparti di di terapia intensiva e subintensiva). È assolutamente necessario - come prevede il decreto-legge in esame - continuare con le misure e gli accorgimenti finora adottati, che si sono dimostrati efficaci, evitando così la necessità di un nuovo *lockdown* nazionale - come invece è accaduto in altri Paesi europei - a partire dalla proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 30 aprile 2021; misura prodromica a qualsiasi altra per la gestione della pandemia. Sono Sono infatti preoccupanti il numero crescente di varianti e la velocità di contagio, che rimane tutt'oggi allarmante. I numeri rilevati nella prima metà di gennaio avevano allarmato gli esperti del CTS, soprattutto in proiezione delle settimane successive, che indicavano un'elevata probabilità di innalzamento dei contagi per quella che sarebbe potuta essere la cosiddetta terza ondata. Sempre in argomento, vorrei ricordare che il precedente Governo è stato più volte fatto oggetto di riconoscimento e portato ad esempio riguardo alla gestione dell'emergenza dovuta al Covid-19 da importanti organizzazioni internazionali,

sono stati introdotti nuovi strumenti di finanziamento, tra cui il più importante è di certo il *recovery plan*, che prevede 750 miliardi di euro per la ripartenza europea. L'Italia potrà avere 209 miliardi, ossia la quota più alta destinata a un singolo Paese dell'Unione europea. il 2020 il precedente Governo ha adottato numerosi provvedimenti per contrastare i pesantissimi effetti negativi sulla salute pubblica e sulle attività economiche del Paese, a seguito delle necessarie misure di contenimento per la per la diffusione del contagio, mettendo in campo complessivamente più di 108 miliardi di euro in termini di indebitamento netto, reperiti attraverso quattro successivi scostamenti di bilancio. A ciò si aggiungono 40 miliardi previsti nella legge di bilancio 2021. Sul tema vorrei inoltre ricordare che, a seguito dell'arrivo della seconda ondata di pandemia nell'ultimo trimestre del 2020, che ha reso necessarie nuove misure per il contenimento del contagio attraverso la restrizione delle attività economiche a livello regionale e comunale, il Governo Conte ha varato - in poco più di un mese - quattro decreti-legge ristori per complessivi 18 miliardi di euro in termini di indebitamento netto, di cui otto finanziati con ulteriore scostamento di bilancio, con un insieme di misure rapide, il più possibile automatiche - tra cui contributi a fondo perduto, sospensione e riduzione di imposte, contributi, versamenti e nuove settimane di cassa integrazione - destinate alle categorie più colpite dalle nuove restrizioni. Era stato previsto anche un quinto decreto-legge ristori per fine gennaio 2021, finanziato attraverso un nuovo scostamento di bilancio, approvato dal Parlamento, di 32 miliardi di euro, ma non è stato possibile emanarlo a causa della crisi di Governo iniziata con le dimissioni dei Ministri di Italia Viva annunciate da Matteo Renzi. Un quinto decreto-legge ristori si sarebbe già dovuto approvare e rendere operativo da tempo, perché nell'ultimo mese vi sono stati innumerevoli passaggi di Regioni e Comuni a scenari di gravità più alta, fino al colore rosso, senza che, a fronte di nuove restrizioni e chiusure delle attività economiche, fossero stati prontamente resi disponibili i conseguenti e necessari ristori. Ho ritenuto di ricordare l'enorme lavoro fatto

da parte dell'AIFA, a partire dal 22 dicembre 2020, possano arrivare nei mesi a venire ed essere somministrate a decine di milioni di cittadini. Nel provvedimento in esame viene introdotta - all'articolo 3 - la piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare - sulla base dei fabbisogni relativi - le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione e relativo tracciamento. Alle Regioni e alle Province autonome sono affidate le diverse fasi di vaccinazione per la prevenzione dell'infezioni da Covid-19, ivi inclusa l'offerta attiva alle categorie di assistiti individuate in base a criteri indicati dal piano strategico dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da Covid, adottato con decreto del Ministro della salute il 2 gennaio 2021. Pertanto, nelle more del decreto-legge in conversione, le Regioni e le Province autonome sono chiamate a svolgere un'importante azione a livello territoriale, nel rispetto delle funzioni loro assegnate dalla Costituzione, nell'abbreviare i tempi per superare questa pandemia e tornare al più presto a quelle che erano le condizioni di vita sociale

figura al penultimo posto tra le Regioni nel numero di vaccinazioni eseguite ogni 100.000 abitanti e al terzultimo posto come rapporto percentuale tra dosi di vaccino consegnate e dosi somministrate, pari al 61 Mi è stato inoltre segnalato che l'Umbria è l'unica Regione che non somministra il vaccino la domenica, nonostante vi sia ancora un 44 per cento di dosi già consegnato e pronto per essere somministrato. Dunque, vorrei anche inviare un'esortazione affinché nella mia Regione

Governo, onorevoli colleghi, prima di addentrarmi nei temi del decreto-legge in esame, proprio in considerazione della diretta rilevanza del provvedimento in discussione, ritengo doveroso porgere i miei migliori auguri al dottor Fabrizio Curcio e al generale Francesco Paolo Figliuolo per gli importanti incarichi che sono stati loro assegnati in questi giorni. *(Applausi)*. Li attende un lavoro difficile, ma che siamo certi svolgeranno al meglio; lavoro per il quale avranno, da parte nostra, piena collaborazione. L'emergenza che stiamo affrontando non accenna a diminuire il suo impeto, ma oggi, a fronteggiarla, trova un Esecutivo a mio avviso più pronto; un Esecutivo che non si lascia sopraffare dalla paura, ma lavora con spirito costruttivo, non si difende ma contrattacca; un Esecutivo che, con una mano, è impegnato a fermare la pandemia, ma, con l'altra, è al tempo stesso proteso a tracciare la strada della ripartenza. Il provvedimento in esame oggi è eredità del vecchio Governo e, come altri provvedimenti del precedente Esecutivo, mostra lo stesso problema, più volte sollevato dal nostro Gruppo parlamentare: soluzioni adottate in ritardo nel tentativo di rincorrere gli eventi; una visione opposta alla nostra, che non può essere efficace se vogliamo proteggere i nostri concittadini e, allo stesso tempo, rilanciare il nostro Paese. Proprio a testimonianza delle considerazioni appena espresse, le nostre proposte emendative al testo erano tese a portare, dal nostro punto di vista, delle migliorie capaci di conferire al provvedimento una portata sicuramente maggiore, con un impatto capace di garantire benefici, tanto immediati quanto futuri. Questo aspetto lo ravvisiamo in maniera preponderante nell'articolo 3 del testo in esame: la disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. chiaro a tutti che, se vogliamo superare e sconfiggere questa pandemia; se vogliamo operare importanti riaperture e gettare basi sempre più solide e tangibili per la ripartenza, questo passa - *in primis* - da una campagna di vaccinazioni seria, importante molto differente da quella che è stata impostata e portata avanti fino ad oggi e che ci vede ancora impegnati a raccogliere dati in un momento nel quale, invece, ci saremmo dovuti ritrovare a vaccinare. Il nostro suggerimento, volto a razionalizzare al massimo i tempi e i costi e a raggiungere risultati immediati, era quello di utilizzare una struttura già esistente come l'Anagrafe nazionale vaccini presso il Ministero della salute, andando a potenziarne e ad adeguarne la relativa dotazione tecnologica applicativa. A nostro avviso, questo avrebbe consentito di dare davvero piena, celere e trasparente attuazione al piano straordinario dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e avrebbe consentito a una struttura, già pronta e implementata come da necessità, di far fronte meglio, prima e con minori costi, a tutte quelle esigenze di supporto, raccordo e comunicazione che l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede in capo alla istituenda piattaforma informativa nazionale. Mi auguro che tale piattaforma operi in modo snello ed efficace e non solo porti al raggiungimento della verifica delle dosi e dei materiali necessari per effettuare le operazioni di vaccinazione, ma possa essere anche efficacemente utilizzata per semplificare la parte burocratica, che rallenta le operazioni di vaccinazione. In particolare, auspico che, al momento della prenotazione *on line*, diventi possibile compilare già il consenso informato e il modulo di anamnesi medica, che attualmente sono compilati su moduli cartacei quando ci si presenta per la vaccinazione, con conseguente rallentamento delle operazioni. È chiaro a tutti che la realtà che viviamo deve suggerirci di preparare e strutturare le nostre istituzioni in modo che nessuna eventuale criticità futura possa trovarci vulnerabili e impreparati come accaduto per la pandemia che stiamo affrontando. È necessario un cambio di marcia. I primi passi sono stati mossi nella direzione tracciata dal presidente Draghi nel suo discorso alle Camere, con la sostituzione operata ai vertici della Protezione civile e della struttura commissariale di emergenza. Ma non possiamo fermarci qui: dobbiamo analizzare gli errori fatti in precedenza e capire che cosa poteva essere fatto meglio, al fine di riuscire a riemergere più velocemente possibile dallo stato emergenziale. Proprio in questa direzione auspico che si muovano le prossime decisioni in materia, perché, se vogliamo far ripartire l'economia, riaprire le attività, permettere agli studenti di frequentare le lezioni non più a distanza, ma dal vivo, dobbiamo prevenire i possibili sviluppi pandemici e giocare in anticipo. A questo riguardo, mi viene in mente il *test* di rilevamento salivare. È di questi giorni la notizia che ricercatori del laboratorio LABION dell'IRCSS-Fondazione Don Gnocchi, in collaborazione con il laboratorio MIND, guidato dalla professoressa Enza Messina, del Dipartimento di informatica sistemistica e comunicazione dell'università di Milano Bicocca, hanno condotto una ricerca che ha portato alla messa a punto di un esame diagnostico per rilevare la presenza del Covid-19 nella saliva dei pazienti: un esame rapido, sicuro, per nulla invasivo, che, grazie a una innovativa tecnica in ambito clinico, è in grado di dare un risultato altamente sensibile e specifico entro pochi minuti e di rivelare anche la gravità della patologia respiratoria intercorsa e il tempo trascorso dall'infezione. La possibilità di effettuare *test* efficaci in poco tempo permetterebbe di eseguire facilmente un numero rilevante di esami e avere dati sull'evoluzione epidemiologica giornaliera, con la conseguente capacità di adottare strategie di contenimento in modo tempestivo e senza ritardo. Inoltre, si avrebbero delle implementazioni della capacità di tracciamento e individuazione iniziale di possibili focolai, ambito nel quale - purtroppo - fino a oggi abbiamo avuto problemi con le conseguenti recrudescenze con le conseguenti recrudescenze a tutti noi note. Una maggiore efficienza nella tracciabilità ci permetterebbe anche di monitorare costantemente il diffondersi delle varianti e individuare più velocemente eventuali nuove forme, con la conseguente possibilità di adottare in anticipo le migliori strategie preventive di cura. A questo riguardo, ho apprezzato che il nuovo Governo si sia prontamente attivato anche per individuare sul nostro territorio le imprese che siano immediatamente in grado di produrre i vaccini già in commercio o che, nel breve periodo, siano in grado di attrezzarsi per la produzione. Personalmente auspico che, pur rispettando gli impegni già presi a livello europeo per la distribuzione dei vaccini, nell'ambito delle strategie preventive si possano vagliare anche strade similari a quelle intraprese da Austria e Danimarca per lo sviluppo di vaccini di seconda generazione capaci di resistere alle varianti del Covid-19. Presidente, mi accingo a concludere facendo mia una frase di Martin Luther King, con l'auspicio che possa aiutare noi tutti nel trovare l'audacia necessaria per riemergere dalla difficoltà che ci ha travolti: «Un giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno». Per il bene dell'Italia e dei suoi cittadini servono coraggio per affrontare il presente e visione per scrivere il futuro. Il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione c'è, coraggioso, audace e fiero di fare la propria parte.

da più di un anno rivolgo la mia attenzione con una certa sofferenza ed è quello della scuola. La scuola non è entrata a sufficienza da subito, ma neanche successivamente, nel dibattito

anche nel rapporto di Save the Children. Certo, si dice che i criteri a cui i governatori dovranno

si lascia in mano ai governatori - e sembra anche ai sindaci - la possibilità di assumere decisioni localistiche. Ho sentito che anche i dirigenti i dirigenti scolastici avranno una certa libertà di scelta, ma così non deve essere perché il diritto all'istruzione è sancito dalla Costituzione e deve essere garantito in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Ma questo non è stato. Chiaramente siamo tutti coscienti - è superfluo anche ripeterlo - che la sicurezza sanitaria è al primo posto,

Sappiamo benissimo però di non avere un'equa distribuzione di questi dati sul territorio nazionale e che il Sud è altamente danneggiato da ciò, anche perché la DAD non è possibile ovunque, in quanto penalizzata dalla mancanza di collegamento alla rete in moltissime parti del territorio nazionale e dal

e si investiranno solo 800 milioni per il trasporto locale, anche se sappiamo che è a causa della carenza del trasporto pubblico locale che le scuole non possono assicurare

Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, le misure contenute nel decreto-legge che oggi andiamo ad approvare recano ulteriori provvedimenti in materia di contenimento e di prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. La *ratio* che guida ancora una volta i provvedimenti e i contenuti deriva sempre dalla necessità di arginare il più possibile la diffusione del virus e la risalita dell'indice dei contagi. Il messaggio chiaro e deciso trasmesso, che deve arrivare ai cittadini, coinvolgendoli in modo attivo in un'adesione convinta e partecipata alle misure adottate, risulta essere sempre quello di rimarcare l'importanza fondamentale dei corretti comportamenti da tenere da parte di tutti, la necessità comunque di sacrifici e di limitazioni, la priorità di preservare in tutti i modi possibili la salute individuale e della collettività, considerandola bene inalienabile, a prescindere dalle complesse problematiche e dalle profonde ripercussioni che ciò comporterà sugli equilibri sociali e sulle attività economiche e commerciali. Casomai occorre considerare che la maggiore difficoltà, come in tutte le cose, è riuscire a ottenere il giusto equilibrio tra la prevenzione sanitaria

e le stesse scuole, aperte o chiuse in maniera disomogenea su tutto il territorio nazionale, in virtù dei provvedimenti attuati dai governatori. Tutte queste ultime strutture rappresentano non solo punti di aggregazione sociale, ma spazi in cui avvengono momenti importanti della crescita culturale globale di una collettività. Tutto ciò si dovrà realizzare, ovviamente, nel rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sociale. Il rapido diffondersi delle varianti del virus su tutto il territorio nazionale non deve e non può essere assolutamente sottovalutato da nessuno. Le diverse varianti, come ormai dimostrato, hanno una maggiore e più alta contagiosità e capacità di diffusione, coinvolgendo rapidamente e progressivamente in particolare le persone più suscettibili della nostra comunità. Non è con la paura e le fobie o, al contrario, con l'incurante ostentazione di sicurezza, né con le parole inutili, che si fa il bene di tutti, ma con i fatti concreti e con i comportamenti responsabili, anche stigmatizzando atteggiamenti inaccettabili e denunciando con forza tutti gli eccessi e gli abusi che cittadini poco responsabili compiono, incuranti dei tanti sacrifici, non solo economici, e delle innumerevoli privazioni, anche affettive, che la stragrande maggioranza della comunità, in maniera responsabile, responsabile, attua ogni giorno e costantemente. La strada maestra per combattere la pandemia, capace di portarci finalmente a vedere la luce in fondo al *tunnel*, è stata già tracciata dal Governo precedente, pur tra le tante difficoltà e alcune criticità legate alla lentezza della macchina burocratica, a una struttura organizzativa farraginosa e agli interventi decisi, spesso in controtendenza, e attuati dai diversi governatori regionali, volte non in sintonia con le direttive governative, cosa questa, peraltro, che ovviamente è consentita dal Titolo V della nostra Costituzione. Fondamentale sarà un migliore coordinamento con le strutture regionali e territoriali: solo una maggiore armonizzazione e un miglior collegamento di tutti gli organismi coinvolti nei processi decisionali permetteranno di ottenere risultati via via più concreti, in tempi più rapidi e sempre più efficaci, nella lotta al coronavirus, che consentiranno di non vanificare gli sforzi e i sacrifici di tanti. Finora abbiamo dovuto rincorrere il virus; ora, grazie alla potente arma del vaccino, che la scienza e la ricerca, con grande sforzo, impegno e competenze, sono riuscite a realizzare, mettendola a disposizione della comunità internazionale, si è riusciti a realizzare un punto fermo ed efficace, capace finalmente di capovolgere i ruoli e di contrastare l'impatto e la violenza del virus sullo stato di salute di tutti noi, soprattutto delle persone più fragili e deboli. Occorre ora fare presto e bene, proseguire e implementare in maniera decisiva la campagna vaccinale, accelerare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale la distribuzione delle dosi vaccinali, razionalizzando la struttura organizzativa e l'utilizzo degli operatori sanitari, permettendo così di raggiungere fasce sempre più ampie della popolazione, nel rispetto delle priorità e delle necessità stabilite. Si tratta della più grande e impegnativa campagna di prevenzione sanitaria mai attuata, non solo nel nostro Paese, ma nel mondo. Più rapida, massiccia e inglobante sarà l'immunizzazione di massa, minore possibilità si darà al virus di mutare e di far sentire i suoi effetti. Mentre sempre più persone si vaccineranno, riuscendo a raggiungere in tal modo percentuali di vaccinati tali da permettere di garantire l'immunità di gregge, è indispensabile per ora ridurre il più possibile la circolazione e la diffusione del virus. Per ottenere ciò, come sappiamo, occorrono l'adesione e la partecipazione di tutti alle misure previste, alle raccomandazioni di protezione individuale e, purtroppo, anche a chiusure temporanee o a un uso contingentato di spazi, strutture strutture e attività che possono facilitare, in modo involontario, ma scientificamente dimostrato, assembramenti o comportamenti che favoriscono la circolazione del virus e la possibilità di contagio. Il ricordo del dolore profondo che ha colpito tutti noi, segnando in maniera indelebile migliaia di famiglie nei sentimenti più intimi per la perdita dei loro cari,

e ad andare avanti, pur nelle difficoltà, nelle rinunce e nei sacrifici, con tanta forza d'animo e spirito di coesione.

nonché provvedimenti mirati, sia in campo sanitario, sia in ambito sociale, economico e ambientale, per poter finalmente ripartire e guardare con più ottimismo al futuro. *(Applausi)*.

ci sono molte zone rosse nel nostro Paese e si teme anche per intere Regioni. Nella mia, il Piemonte, ci sono 22 Comuni in zona rossa, tra cui uno a settanta metri da casa mia,

di tenere conto delle zone dichiarate rosse, con tutte le limitazioni che hanno, per privilegiarle e consentire loro una qualche forma di precedenza e priorità nella campagna vaccinale. Questa è una richiesta che viene veramente dal territorio e dai sindaci che gestiscono, con grande difficoltà, situazioni difficili.

del Consiglio dei ministri. Il decreto-legge ha il grosso vantaggio di essere previsto dalla Costituzione e vi sono un vaglio preventivo del Presidente della Repubblica e un controllo immediato del Parlamento, con la possibilità

il Governo Conte aveva usato e che il Governo Draghi ha usato proprio il 22 febbraio scorso. Ora siamo tornati all'altro strumento. Mi chiedo perché e auspico che si ritorni a utilizzare gli strumenti propri, previsti dalla Costituzione, come abbiamo chiesto tante volte in vari atti da noi presentati.

sono felice di intervenire oggi, in questa settimana che è un nuovo inizio, perché finalmente la nostra squadra di Governo è al completo. Faccio ovviamente il mio in bocca al lupo ai colleghi della Lega che sono entrati nella squadra dei Sottosegretari, ma anche a tutti gli altri, perché se vogliamo davvero essere un Governo di unità nazionale dobbiamo imparare, dopo un periodo difficile di scontri, anche molto accesi, a lavorare bene insieme e con rispetto reciproco. Il lavoro della 1a Commissione è stato un banco di prova interessante, perché ci siamo ritrovati per la prima volta - cosa di cui ringrazio il sottosegretario Malpezzi,

quindi aria nuova, con persone di tutto rispetto, che hanno già dimostrato nel loro settore di saper lavorare bene, quindi ci auguriamo che anche per la parte più tecnica della gestione della pandemia ci sia un nuovo corso.

stanca, perché, anche se all'inizio si prospettava uno scenario che non comprendevamo e non conoscevamo, c'era la speranza che finisse in fretta,

la frase ricorrente e generalizzata per tutto l'arco costituzionale è: mettete misure restrittive, passa un Governo e ne arriva un altro, ma voi lo stipendio fisso - e anche abbastanza importante - lo avete, quindi cosa vi importa se noi siamo a casa e non abbiamo da mangiare?

vero, nel senso che nessuno prende le decisioni alla leggera e da sindaco lo so, avendo gestito la fase più critica dell'emergenza Dobbiamo spiegare alla gente la bontà delle decisioni e, a volte, anche del modo in cui si comunicano. Mi pare che il *premier* Draghi abbia avviato anche a tal proposito un nuovo metodo, forse meno da protagonista, ma più concreto e veloce.

Servono anche in questo periodo più controlli sul territorio, perché, come diceva il collega Malan, i sindaci sono molto preoccupati e hanno bisogno di sostegno e di aiuti. Vi faccio solo un esempio: stiamo aspettando il decreto attuativo per dare i contributi per l'assunzione di personale a tempo determinato all'interno dei Comuni per gestire il superbonus. Sembra che non c'entri niente con la pandemia, ma in realtà c'entra, eccome, perché gli uffici tecnici sono oberati e l'ufficio tecnico solitamente segue anche il centro operativo comunale (COC) di protezione civile. Pertanto, più peggiora l'emergenza, più l'ufficio tecnico si deve occupare di questioni sanitarie e meno tempo a preoccuparsi di tutto il resto del lavoro. Abbiamo bisogno di aiuti rapidi e concreti per le nostre attività e anche per le nostre famiglie. Mi pare di intuire anche che il meccanismo

poi la questione importante dei vaccini. In Lombardia stiamo già dando un occhio di riguardo alle zone più colpite: partendo partendo dai Comuni del Bresciano, ci si è allargati alla fascia cuscinetto di quelli del Bergamasco e oggi partono le adesioni per la campagna vaccinale nelle scuole; pertanto, grazie anche alla Regione Lombardia, alle zone più colpite, proprio per arginare questo contagio che sta notevolmente aumentando, con una velocità preoccupante soprattutto a causa delle nuove varianti. Con gli

per fare la spesa e quant'altro). Sempre nell'ottica, da una parte, di organizzare il lavoro dei Comuni e, dall'altra, di non creare problemi ai cittadini, trovare un metodo - e so che se ne è parlato anche al Governo, ma non era questo il momento per sistemare la questione - per

ma poi arriveremo a un punto in cui tutto scadrà esattamente lo stesso giorno e bisognerà capire come fare, perché la gente dovrà fare file chilometriche per avere i documenti. Occorre quindi cominciare a pensare a una dilazione, prendendo magari spunto dai documenti che sono scaduti prima, perché queste proroghe vanno avanti da più di un anno, e cominciare a evadere, in quanto i nostri Comuni comunque non sono fermi, non è che non hanno più fatto carte d'identità;

si dovessero chiudere ancora le scuole: penso alle zone rosse, ma anche ai nuovi criteri adottati sulla percentuale di contagi anche in quelle arancioni e gialle. Dobbiamo quindi trovare velocemente una soluzione a questo problema, sia con aiuti economici sia con *bonus baby sitter* o quant'altro, ma facciamo in modo che la gente e le nostre famiglie non si sentano abbandonate. ringraziamento per la collaborazione che c'è stata in questi giorni; sono felice di poter dare finalmente un contributo fattivo anche all'interno di questo nuovo Governo. In questa fase così grave, grave, da bergamasca e da sindaco, non posso che mandare un abbraccio alla mia gente e ai miei colleghi, in particolare di Bergamo, perché siamo molto preoccupati di questo nuovo periodo che ci attende.

Presidente, con il decreto-legge n. 2 del 2021, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza sanitaria da coronavirus e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, il Consiglio dei ministri ha dichiarato per ulteriori tre mesi, e fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza nazionale, estendendo l'applicabilità delle misure restrittive già previste dal decreto-legge n. 19 del 2020, nonché delle ulteriori misure circa spostamenti, riunioni e svolgimento delle attività economiche di cui al decreto-legge n. 33 del 2020. Il secondo Governo Conte è finito ed è iniziato un Governo nuovo, quello del Presidente, perché il professor Draghi è stato scelto direttamente dal presidente Mattarella e non dalle forze politiche in Parlamento. Tuttavia, la pandemia resta e così le sue gravissime conseguenze sul piano socio-economico. Ecco quindi che l'agenda politica continua a essere dettata dal virus e le misure restrittive della libertà di spostamento dei cittadini continuano ad essere determinanti al fine del contenimento della diffusione del contagio. il provvedimento che oggi ci accingiamo ad approvare disciplina il divieto di spostamento tra Regioni fino al 15 febbraio, misura in realtà già ulteriormente prorogata fino al 27 su tutto il territorio nazionale dal Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2021, salvi, naturalmente, gli spostamenti per comprovate esigenze di lavoro, salute e necessità, nonché il divieto di spostamento all'interno della stessa Regione e Provincia, con i limiti e le condizioni previsti per gli spostamenti presso abitazioni private tra le ore 5 e le ore 22 in zona gialla e all'interno dello stesso Comune in zona arancione, nel limite di due persone, oltre ai figli minori di anni quattordici e disabili. Si tratta quindi di un decreto che adotta un criterio di mappatura dell'Italia in diverse zone colorate a seconda del coefficiente RT, dunque un criterio flessibile, in quanto prevede una gradualità di limitazioni a seconda che la Regione interessata sia appunto gialla, arancione, rossa o bianca (come è oggi la Sardegna), e che fa superare il più pesante e generalizzato *lockdown* totale, che abbiamo conosciuto nei primi mesi della pandemia e che, se protratto ulteriormente, avrebbe pregiudicato più gravemente la situazione socio-economica del Paese. Vediamo infatti che ancora oggi i dati attuali del contagio non sono rassicuranti, perché in 12 Regioni non scendono, ma aumentano i casi positivi, in tre l'occupazione dei posti letto in ospedale supera la soglia del 40 per cento in area medica in cinque quella del 30 per cento delle terapie intensive. L'indice RT, infatti, è appena sotto l'1 e la cosa che più preoccupa i virologi è la diffusione della variante inglese al Covid-19, presente purtroppo in 14 Regioni delle 16 prese in considerazione. In ordine alla vaccinazione, il decreto-legge che oggi intendiamo intendiamo approvare definisce alcuni profili dell'attività di vaccinazione già oggetto di un apposito piano strategico nazionale, prevedendo l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale predisposta e gestita dal commissario straordinario. Essa è destinata ad agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali e a svolgere le operazioni di prenotazione e registrazione delle vaccinazioni, laddove il sistema informativo vaccinale delle Regioni non risulti adeguato. tuttavia, la campagna di vaccinazione procede a rilento, perché non vi è un adeguato piano strategico vaccinale regionale. Incombe la burocrazia, mancano i centri vaccinali organizzati. Penso in particolare alla mia Regione, la Sardegna, che risulta al terzultimo posto in Italia per percentuale di popolazione che ha completato il ciclo: circa l'1,59 per cento, laddove la media nazionale è del 2,18. La Giunta regionale ha sponsorizzato una piattaforma CUP *web* per le prenotazioni mai attivata, il piano vaccinale per gli anziani *over* 80 è ancora fermo, salvo una piccola cerchia nel Sud della Anche la vaccinazione dei docenti è a rilento e terminerà, purtroppo, ad anno scolastico finito. Lo stesso accade per le categorie fragili: penso ai 500 non vedenti che avrebbero dovuto essere vaccinati a febbraio e che penso ai migranti; per non parlare poi delle Forze dell'ordine, una delle categorie più esposte al contagio, che lamentano anche dubbi sull'efficacia del farmaco. È notizia solo di qualche giorno fa il coinvolgimento dei medici di base in questa campagna di vaccinazione, grazie a un accordo Governo-Regione, con la conseguenza di dare un po' più di respiro agli altri comparti sanitari. Anche loro attendono le dosi per partire, però, laddove ci sono i medici di medicina generale. Anche sotto questo profilo non posso non segnalare la grave assenza dei medici di famiglia in tutto il territorio del nuorese, denunciata dai nostri sindaci. Penso in particolare all'ordinanza di qualche settimana fa del sindaco di Oniferi, in provincia di Nuoro, che testualmente vietava ai cittadini di ammalarsi, soprattutto di Covid. Occorre pertanto che il Governo intervenga al più presto sulle Regioni, al fine di monitorare ed eventualmente intervenire, laddove le amministrazioni regionali arranchino. Anche il comparto giustizia ha bisogno di ripartire a pieno regime e in sicurezza. All'arretrato consolidato in molti anni si è aggiunto quello dell'anno di Covid; non possiamo permetterci di ledere ulteriormente diritti e funzioni previsti dalla Costituzione. Per questo anche gli avvocati, e non solo i magistrati, debbono essere inseriti tra le categorie da vaccinare in via prioritaria in tutte le Regioni, cosa che ancora non è accaduta. Sono loro, insieme ai giudici togati e onorari, la categoria che nei tribunali ha pagato di più le conseguenze della pandemia in termini economici e di difficoltà a svolgere il lavoro. Anche nelle carceri bisogna accelerare, per tutelare sia i detenuti sia gli agenti di Polizia penitenziaria. In questi mesi abbiamo potuto riscontrare enormi difficoltà nel garantire il distanziamento sociale nelle carceri e nei tribunali e pertanto abbiamo visto quanto sia importante investire nell'edilizia carceraria e penitenziaria, per garantire a tutti i cittadini un efficiente sistema giustizia. Tornando al provvedimento che oggi siamo chiamati a votare, il sistema sanzionatorio previsto è puntuale e articolato; esso mira a rafforzare l'osservanza delle misure in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza sanitaria, al fine di evitare quanto già accaduto in altri Paesi. Pensiamo agli Stati Uniti, dove il numero dei morti è superiore a quello totale delle vittime della Prima e della Seconda guerra mondiale e della guerra in Vietnam. Il nostro intervento legislativo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento a tutti ormai note venga punito secondo le disposizioni contenute nei decreti-legge nn. 19 e 33 del 2020, ossia la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 400 a 1.000 euro. Non si applica invece più la sanzione penale di cui all'articolo 650 del codice penale. Se il mancato rispetto avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, la predetta sanzione è aumentata fino a un terzo, mentre nell'ipotesi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa produttiva o commerciale, viene altresì applicata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio dell'attività da cinque a trenta Nell'ipotesi specifica dell'inosservanza della quarantena, la sanzione invece è quella dell'arresto fino a diciotto Concludo, signor Presidente. Tale sistema sanzionatorio non ci esime dal richiamo al senso di responsabilità personale, attraverso l'uso delle mascherine e il distanziamento sociale, che mai come ora, nella drammatica emergenza determinata dalla pandemia, si traduce in un senso di responsabilità collettiva. La strada dell'unità e della responsabilità rimane l'unica possibile nella guerra a questo nemico invisibile, al fine di garantire a tutti, soprattutto ai nostri figli, una vita normale e un futuro libero da impedimenti e restrizioni. Ringrazio l'Assemblea tutta.

Una recente sentenza del TAR del Lazio ha detto che il Governo non può più chiudere le scuole senza dati specifici. L'*escamotage* di collegare la chiusura delle scuole al tasso generale dei contagi pare non sia sufficiente. Dovremmo quindi sapere quanti sono i casi negli istituti e soprattutto i doppi casi nelle singole classi, per capire la trasmissibilità. È indifferibile, dunque, che l'Italia disponga di una propria rilevazione, di respiro nazionale e con carattere multicentrico, sui determinanti sociali dell'infezione da SARS-CoV-2, attraverso la creazione di una rete di collaborazione tra Istituto superiore di sanità, Regioni e altre istituzioni del mondo la ricerca, come le università. Come evidenziato di recente dai professori Alleva e Zuliani, i dati finora comunicati non sono utili per capire come stia evolvendo il Covid-19; per esempio, si rileva la discrepanza tra i risultati dati dai *test* rapidi e quelli dati dagli altri esami diagnostici. In questa incertezza, il dato sul tasso generale di positività risulta poco attendibile; stesso dicasi per i ricoveri e per i dati sulla mortalità, che, a giudizio dei due statistici, è sottostimata. Quanto al mondo dell'istruzione, appaiono tanto più necessarie una maggiore trasparenza ed efficienza nella rilevazione e nella comunicazione dei dati, come rilevato da un'associazione di 300 professori universitari, che hanno chiesto l'accesso ai dati per capire come vengono stabiliti i colori delle Regioni. Finora questa richiesta non ha avuto risposta, con il risultato che anche questa controversia è finita nelle mani dal TAR. Non è possibile, a distanza di quasi dodici mesi dall'inizio dell'epidemia, che le principali misure di sanità pubblica siano ancora prevalentemente basate sul principio di precauzione. L'Italia è rimasta una delle poche Nazioni sviluppate che, allontanandosi dalle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, utilizza ancora il criterio dell'accertamento diagnostico attraverso il tampone negativo per la dichiarazione di guarigione, previsto dalla circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020. L'Organizzazione mondiale della sanità e diverse Nazioni, come Stati Uniti, Francia e Belgio, si erano già espresse in merito, delineando in diversi documenti tecnici come tale criterio sia da ritenersi obsoleto e dannoso, determinando un fenomeno di sovraccarico di lavoro anche per il Servizio sanitario nazionale. Questo dato, già da solo, determina un'importante adulterazione delle nostre cifre epidemiologiche nazionali e, di conseguenza, regionali. Inoltre, il sistema di classificazione del rischio è basato principalmente sul cosiddetto indice RT, che, sulla base delle evidenze più recenti, sembra essere un indice non eccessivamente precoce nel predire il rischio epidemico (presenta, ad esempio, un ritardo medio di una settimana rispetto alle variazioni percentuali). Pertanto, i parametri ad oggi utilizzati fanno correre alla Nazione il rischio di inseguire la curva epidemica nel delineare le azioni della sanità pubblica, piuttosto che prevenire l'epidemia. Il disegno di legge in esame prevede anche la creazione di una infrastruttura tecnologica a supporto delle azioni del commissario per l'emergenza, per la distribuzione alle Regioni di vaccini e presidi funzionali al processo di vaccinazione, che sia interoperativa con l'Anagrafe nazionale dei vaccini. Tale piattaforma dovrebbe avere anche una funzione sussidiaria rispetto alle anagrafi vaccinali regionali, supportando azioni quali la prenotazione, la registrazione delle vaccinazioni effettuate e la certificazione dell'avvenuta vaccinazione. Su quest'ultimo punto è indifferibile intervenire delineando i requisiti minimi della certificazione di avvenuta vaccinazione, in relazione anche ai possibili utilizzi che questa certificazione potrà avere nel futuro prossimo. Le informazioni aggregate presenti sulla piattaforma sono accessibili al Ministero della salute, all'Agenzia italiana del farmaco e all'Istituto superiore di sanità. Per le attività di valutazione di immunogenicità, invece, i dati disaggregati e nominativi sono resi disponibili solo per l'Istituto superiore di sanità. Questa previsione andrebbe aggiornata, come hanno riferito nelle audizioni alcuni illustri docenti, conferendo la visibilità dei dati disaggregati anche all'Agenzia italiana del farmaco, al fine di consentire alla stessa un migliore esercizio delle attività di farmacovigilanza. In ordine alle previsioni del disegno di legge, devo innanzitutto evidenziare come le originali previsioni del Piano strategico per le vaccinazioni in materia di scadenziario delle popolazioni *target* dell'intervento vaccinale dovranno essere con urgenza riviste in relazione all'effettiva disponibilità di vaccinazioni, nonché alle limitazioni previste nell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino prodotto dalla ditta AstraZeneca. È inevitabile che la disponibilità di dosi di un vaccino idoneo all'immunizzazione di soggetti al di sotto dei cinquantacinque anni di età porti all'opportunità di anticipare le vaccinazioni di categorie di giovani adulti lavoratori. Nell'impossibilità di una protezione diretta dei soggetti più anziani e fragili, dovrà essere percorsa la strada dell'immunizzazione di larghe fasce di popolazione a maggior rischio di contrarre l'infezione, al fine di raggiungere, almeno parzialmente, l'obiettivo di incidere sulla circolazione del virus, andando a modificare, attraverso questo obiettivo, il dato di morbilità e mortalità. In quest'ambito andranno privilegiate scuole e università, in quanto il danno principale che la pandemia sta creando al nostro Paese è proprio quello relativo alla formazione delle nuove generazioni. Gli effetti di questo danno condizioneranno più degli altri la possibilità di sviluppo dell'Italia nei prossimi trenta, Non è il caso di ribadire che la pandemia continua ad avere ripercussioni significative sulla vita reale delle persone, delle famiglie e degli operatori economici. Nella mia Regione, appena dichiarata zona rossa, la questione si è spostata dal piano tecnico-scientifico a quello politico, con una *querelle* tra il Presidente della Regione e le singole amministrazioni. Ciò non sembra essere utile al confronto tra i diversi attori in campo chiamati a gestire, ciascuno per la propria parte, l'emergenza sanitaria. La dichiarazione della Basilicata come zona rossa non è stata una scelta della Regione, ma esclusiva del Ministero alla salute, e la decisione è fondata su parametri che, per quanto oggettivi, non tengono conto della specificità dei territori.

l'integrazione del Comitato tecnico-scientifico, che ci ha accompagnato in quest'anno di epidemia, con professionalità diverse: esperti di analisi dei dati fisici, matematici, microbiologi. Si sente il bisogno, in questo tempo, di anticipare il virus e non più di inseguirlo, e per raggiungere tale obiettivo occorre la contaminazione di competenze diverse. In Italia ne abbiamo tante e di eccellenza, dunque facciamole lavorare per noi. Aggiungo che abbiamo presentato a questo provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 2, a cui si è aggiunto il decreto-legge n. 15, un subemendamento per la costituzione di un osservatorio del dato epidemiologico, di un'analisi quotidiana dell'evoluzione dei contagi da Covid-19, in modo da offrire pareri sulle misure da adottare relativamente a chiusure limitate, come ad esempio avvenuto a Perugia e per l'Alto Adige, e come sta succedendo in queste ore per la provincia di Bologna. Mi auguro che questa proposta, bocciata in questo provvedimento, trovi accoglienza in uno successivo, perché la riteniamo fondamentale. È giusto aver codificato le Regioni con i colori che indicano il tasso di rischio di contagio, ma risulta fondamentale la messa a disposizione di dati semplici, a livello provinciale e comunale, per decidere velocemente *lockdown* locali. Molte Regioni stanno andando in tale direzione in queste ore, ma è fondamentale un sistema di raccolta, monitoraggio e impatto delle misure quanto più possibile omogeneo a livello nazionale, e che non si basi su informazioni datate di otto, dieci giorni. La velocità esponenziale di crescita dei contagiati da Covid, soprattutto in alcune zone, ci obbliga a un cambio di passo nel prendere decisioni repentine e precise. Immagino interventi mirati su singoli territori per risollevare e guarire l'intera nostra Nazione, facendo leva ancora una volta sul senso di responsabilità dei nostri concittadini, tante volte richiamato in questi mesi. che nel nuovo DPCM firmato dal presidente Draghi ci sia la costituzione di un tavolo tecnico di confronto per la revisione o l'aggiornamento di ventuno parametri per la valutazione del rischio epidemiologico. Anche qui ci auguriamo semplificazione dei parametri. Nel provvedimento in esame ci sono norme importanti sui sistemi informativi funzionali all'alimentazione del piano strategico dei vaccini e all'anagrafe vaccinale, e le Regioni devono collaborare per fornire questi dati. Credo che in Italia ci sia una sorta di maledizione delle banche dati. Mettere in comune i dati è un bene pubblico ed è il più alto indice di di misurazione del grado di democrazia di un Paese. Occorre dare una forte accelerata e raddrizzata al piano vaccinale per questo esprimiamo viva soddisfazione per la nomina del dottor Fabrizio Curcio a capo della Protezione civile e del generale Paolo Figliuolo quale nuovo commissario per l'emergenza Covid, ai quali auguriamo buon lavoro. Pensare di poter impiegare le risorse umane e strumentali della Protezione civile e l'organizzazione logistica dell'Esercito tranquillizza. La Commissione igiene e sanità che mi onoro di presiedere ha deciso ieri di procedere a un affare assegnato sui vaccini per arrivare a un atto di indirizzo, affrontando soprattutto le implicazioni etiche, di ricerca, di scelta delle dosi e disponibilità della produzione in rapporto alle scelte europee.

ha ricordato ancora una volta di prevedere la precedenza per tutte le malattie rare e le patologie gravi e per le persone con disabilità e i loro *caregiver*. Non si possono più tollerare differenze così profonde tra Regioni; il diritto alla cura, soprattutto dei più fragili, è un diritto costituzionalmente garantito. Dobbiamo essere trasparenti tra di noi in questa fase e con i cittadini. Siamo in un momento delicato dell'epidemia, con le varianti che incombono, i vaccini a rilento, un virus nemmeno tramortito (ma solo per qualche settimana stordito tanto da essere in grado di acquisire difese e variazioni), senza vaccinazioni estese, tamponi diffusi, aggiornamenti epidemiologici statistici quotidiani, pochissima assistenza domiciliare, per la quale occorrerebbe (ma non si è fatto finora) un organismo che ne protocolli le cure. Rischiamo così di dover subire il virus prima di controllarne la convivenza; ma bisogna allontanarsi velocemente dal guado per evitare di combattere con un braccio legato dietro la schiena, come avvenuto in Vietnam dove, per mancanza di mezzi e di una strategia, il conflitto fu caratterizzato da una continua guerriglia e dalla visione alla TV dei *marine* feriti. Tralasciando i valori etici di moralità delle guerre, il paragone calza a pennello, a mio avviso; per questo è necessaria una chiamata alle armi del sentimento di un popolo, ripartendo con le energie migliori della Protezione civile, delle Forze armate, del personale socio-sanitario, di professionalità diverse, dei luoghi di lavoro, in un contesto di ordine e semplificazione nel legiferare, di sostegno alle attività economiche e all'occupazione di un rinnovato rapporto di collaborazione tra Stato e Regioni, ma con una fortissima guida centrale. Come ricorda la recente sentenza della Corte costituzionale, spetta allo Stato determinare le misure contro una pandemia diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato a titolo di profilassi internazionale. a mio avviso, ce la faremo, Presidente, onorevoli colleghi; l'Italia è stato il primo Paese in Europa a precipitare nell'epidemia, impieghiamo tutte le nostre forze per essere il Paese modello per l'uscita da essa. Ora abbiamo tutte le carte in regola.

membri del Governo, colleghi, è sicuramente un momento estremamente drammatico; dobbiamo renderci conto che siamo in guerra contro un nemico invisibile. Per poterlo battere dobbiamo mettere in campo ogni strumento che l'Italia e l'Europa hanno a disposizione in questa fase. Plaudo al piglio del Governo, in particolare del

possiamo intraprendere una strada che sarà fatta di organizzazione, tempestività negli interventi, disciplina nelle azioni. Vedete, colleghi, quando si presenta un problema la prima cosa da realizzare è capire cosa avviene, decidere e agire. L'esempio che abbiamo avuto, un esempio di grande visione, è quello del presidente israeliano Netanyahu, che in pochissime ore ha dato avvio a un programma

Siamo disposti anche a pagarli di più. Quanto costano? Costano 15 o 20 euro? Noi li paghiamo 30 euro. Nella stessa giornata, la sera, il presidente Netanyahu ha fatto un bonifico, attingendo ai fondi dell'esercito israeliano, e ha pagato immediatamente i vaccini, senza rateizzare. La mattina

guardando in faccia la realtà, perché la politica è questo. Guardando in faccia la realtà, dobbiamo dire che il momento è drammatico. Guardiamoci intorno. Voglio fare tre osservazioni, rapidamente. La prima: possibile che dobbiamo indirizzarci solamente nei confronti di un solo vaccino? C'è il vaccino della Johnson & Johnson, c'è il Sinovac. In particolare, c'è lo Sputnik, che è un vaccino a vettore virale e non mRNA messaggero e questo è molto importante. Hanno iniziato ad effettuare le vaccinazioni a San Marino, dove si registrano buoni risultati. Sembra sia un vaccino che dà risultati al 90

e si guardi in faccia alla realtà delle cose. Il presidente Draghi ha parlato di autonomia strategica dell'Europa. È un elemento essenziale che ci consentirebbe, anche come Europa, di guardarci intorno e di poter fare questi approvvigionamenti. Voglio ricordare che il 28 gennaio dell'anno scorso fui io a presentare per primo una interrogazione dove evidenziavo cosa sarebbe accaduto in conseguenza della pandemia. Ora dico questo: c'è un altro farmaco, sul quale ho presentato tre interrogazioni, che si chiama Parvulan, è un amplificatore delle difese immunitarie dell'organismo

di quelle zone e anche dell'Italia intera. È necessario, quindi, procedere con operazioni di controllo dei traffici migratori. Dobbiamo farla finita, una volta per tutte, con queste organizzazioni criminali, che sono un bandito appostato sulle strade della civiltà, anche

guardando in faccia il primo problema, dobbiamo assolutamente prendere in mano la situazione e dare risposte concrete, anche con controlli navali e respingimenti.

ci dispiace dover constatare oggi che non c'è stato un cambio di passo con questo nuovo Governo.

Soprattutto ci dispiace vedere molti colleghi, che hanno sempre discusso in maniera anche molto accesa e vivace l'uso del DPCM, i quali invece oggi tacciono

Noi riteniamo che questo strumento sia illegittimo, oltre che anticostituzionale e ci dispiace soprattutto per coloro che

Ricordo che il 90 per cento dei lavoratori e degli studenti si sposta sui treni regionali. Non credo che qualcuno di voi sia mai andato a vedere o abbia mai preso un treno regionale

quella famosa luce in fondo al tunnel. Se infatti non mettiamo al riparo le categorie più fragili, gli *over* ottanta e coloro che hanno delle patologie, come facciamo a uscire dalla pandemia? Capisco che in tale situazione le risposte più facili siano quelle delle chiusure; certo, si potrebbe dire di chiudere tutto. È ovvio che se chiudiamo tutta la nostra Nazione probabilmente il virus smetterà di correre, ma non è questa la situazione. Oggi infatti non siamo più nell'emergenza che, come dice il vocabolario della lingua italiana, è un atto improvviso, per il quale nessuno di noi può essere preparato perché è appunto un'emergenza.

lo stato di normalità nella quale noi umani dovremo imparare a convivere, ma penso che saremo tutti d'accordo nell'affermare che questa situazione non potrà mutare nei prossimi quindici giorni. allora per quale ragione devono essere sempre le stesse categorie a pagare il prezzo più alto, perché sono sempre le stesse categorie che, oltre a pagare il prezzo più alto, sono anche quelle più dileggiate, prese in giro,

affollati. Come mai ieri, quando c'era la possibilità non di parole, ma di fatti concreti, il nostro emendamento in Commissione è stato bocciato? In conclusione, Presidente, dico che gli italiani sono stufi delle parole,

vi consiglierei di usarlo per un piano vaccinale, allora in quel caso, financo noi di Fratelli d'Italia,

darsi da fare. Noi accogliamo finalmente il cambio, che avevamo chiesto da tanto tempo, e la cacciata di Arcuri, con l'arrivo di una persona sicuramente competente e capace, come il generale Figliuolo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi abbiamo in esame reca alcune misure in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica, che ancora oggi non molla la presa, e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

molto prese in considerazione, perché l'epidemia, come detto, sta purtroppo avanzando in maniera preponderante. Quindi, rispetto al provvedimento in esame, prendiamo atto - lo dico ai colleghi che prima hanno parlato molto più del DPCM, che del decreto che stiamo convertendo in legge

3, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, istituisce una piattaforma informativa nazionale per agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione e il relativo tracciamento. Questa piattaforma, come abbiamo detto, è

il Ministero degli affari regionali e le autonomie, informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sullo stato di attuazione del Piano strategico vaccinale, che già c'è da tempo, ma è in corso di modifica. modifica. Le diverse fasi delle vaccinazioni sono affidate quindi alle Regioni e alle Province autonome, che si avvalgono dei propri sistemi informativi vaccinali in qualità di titolari del trattamento. Tuttavia, qualora il sistema informativo vaccinale di una Regione o di una Provincia autonoma non risulti adeguato, su istanza del medesimo ente la piattaforma esegue, in regime di sussidiarietà, come previsto tra l'altro dall'articolo 120 della nostra Costituzione, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni e di registrazione delle somministrazioni dei vaccini. viene fatto in maniera sussidiaria attraverso una piattaforma nazionale che qui viene istituita. A parole tutto bene, ma purtroppo non è così

Ma qui sorgono i primi problemi e ce ne sono due molto importanti: il primo è quello che le Regioni avrebbero dovuto già ottemperare da tempo alla previsione di raccogliere dati certi sulle persone: i soggetti vaccinati, i soggetti da sottoporre a vaccinazione, i soggetti immunizzati i soggetti per i quali le vaccinazioni possono essere omesse o differite; in caso di accertato pericolo per la salute anche la non vaccinazione, perché ci sono dei soggetti fragili, come gli immunodepressi, che non si possono vaccinare; le dosi e i tempi di somministrazione e gli eventuali effetti indesiderati. Tutto questo era già previsto e nel 2019 sono stati messi

con le Regioni e con i territori passo passo quello che si deve fare, perché i territori sono i primi a pagarne le conseguenze. Quindi è giustissimo, per quanto riguarda le chiusure, condividere con le Regioni le decisioni, ma le Regioni devono ottemperare alle normative di legge nazionali. Credo che il famoso conflitto Stato-Regioni debba essere risolto più che mai adesso, proprio perché

Soprattutto in tema di vaccini, abbiamo delle Regioni che hanno i vaccini pronti, ma non hanno i vaccinatori. Abbiamo delle Regioni che hanno i vaccinatori pronti, ma mancano le dosi.

cerchino di risolvere questo problema, perché i cittadini hanno bisogno di essere trattati in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Non è possibile che ci siano alcune categorie protette che non sono ancora state vaccinate, mentre in altre Regioni hanno già vaccinato anche i più fragili, i disabili e quelli nelle RSA. L'altro tema non meno importante che devo assolutamente citare sono i vaccini. La priorità assoluta è avere i vaccini. Le dosi che ci spettano come Paese Italia devono arrivare. La ricerca è stata portata avanti grazie ai fondi pubblici e le aziende devono restituire alla collettività. collettività. Non c'è brevetto che tenga; il vaccino deve essere un bene comune e deve essere dato a tutti. Noi i fondi pubblici li abbiamo spesi; che le aziende facciano un passo avanti. PRESIDENTE. Presidente, colleghi, constato con una certa preoccupazione l'incapacità di questo Parlamento di farsi carico di prendere in mano le sorti del Paese. Da un lato, non vedo alcuna reazione nei confronti del fallimento che l'Europa sta dimostrando nei confronti delle esigenze Non vedo reazioni in relazione all'assoluta mancanza di informazioni circa i contratti e le clausole contrattuali con le aziende farmaceutiche. Non sappiamo quant'è il prezzo dei vaccini; non sappiamo quali sono le clausole di distribuzione e le clausole di responsabilità per le mancate forniture. Eppure non vedo da parte vostra e nostra una reazione e richieste di chiarimenti su questi temi, che hanno delle ricadute evidenti e concrete sui nostri cittadini. Dall'altro, vedo una grande confusione e noto - come qualcuno di voi, invece, ha correttamente rilevato - che si sovrappongono delle fonti eterogenee (alcune non previste dalla Costituzione) che creano l'effetto delle grida manzoniane: decreti-legge convertiti mettendoci dentro anche parti di DPCM precedentemente in vigore; decreti che si susseguono alla velocità della luce non dando il tempo neppure agli addetti ai lavori di comprendere bene qual è il susseguirsi di queste fonti normative. Tutto ciò comporta una grande confusione per i cittadini e il fatto che gli stessi operatori, anche coloro che dovrebbero vigilare sul rispetto di queste norme, non hanno le idee chiare. La conseguenza di tutto ciò è sotto gli occhi di tutti: si hanno idee e linee generali, ma ciascuno le applica a modo suo. Come spesso avviene in Italia, coloro che sono rigorosi

Un caso abbastanza palese è dato proprio dal decreto-legge che dobbiamo convertire oggi, il primo decreto-legge che ha avuto un'importante modifica con un emendamento saliente da parte del Governo dei migliori e che, però, è completamente in continuità con il Governo dei peggiori in quanto a comprensibilità del testo. Faccio un solo esempio concreto. Si dice che fino al 27 marzo è consentita nella zona gialla in ambito regionale e nella zona arancione in abito comunale lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata. Ma se non è abitata? Lo stesso *dossier* del Senato dice a chiare lettere che c'è un vuoto e, cioè, non si norma in nessun caso la possibilità di spostamento nelle seconde case o dalle seconde case. Lo dice chiaro. È stato dimenticato e si fa riferimento alle FAQ, ovvero alle risposte alle domande frequenti pubblicate

dei rappresentanti dei cittadini, cioè del Parlamento, ma a delle risposte pubblicate su dei siti Internet. Tali risposte, che non si sa da prendono il posto della riserva di legge che invece la Costituzione vorrebbe fosse a presidio delle libertà personali. Il risultato è abnorme, paradossale; non c'è discussione su temi fondamentali. Infatti, se è evidente che il diritto alla salute è preminente e importantissimo, è anche chiaro che va bilanciato con tutti gli altri interessi, con le libertà personali, col diritto allo studio, col diritto a poter esercitare le attività economiche. Pertanto, questo bilanciamento che dovremmo trovare noi in realtà sta scivolando in una sorta di ratifica, da un lato, su decisioni prese per quanto riguarda i livelli vaccinali, gli acquisti e quindi le ricadute concrete, sul livello europeo, che noi non mettiamo in discussione e sul quale non vigiliamo; dall'altro lato, sul livello governativo. In questo modo noi apprendiamo, senza senza nessuna particolare discussione, che nelle zone rosse le scuole dovranno essere completamente chiuse, invece nelle altre zone sarà rimessa alla discrezionalità delle Regioni se tenerle aperte o chiuse. Anche questo merita una discussione, perché non è affatto scontato che a livello regionale ci possano essere delle decisioni che penalizzano i nostri ragazzi; i giorni di scuola che verranno persi e che sono già stati persi si ripercuoteranno in maniera drammatica sull'educazione e sulla psiche di queste generazioni, che hanno già delle limitazioni negative sullo sport e sulla loro socialità; togliere loro anche il momento didattico della scuola in presenza, secondo me non dovrebbe essere accettato nel silenzio del Parlamento.

piuttosto far rispettare tutti quei protocolli, anche a costo di investire molto ad esempio sulla mobilità degli alunni e su tutti gli spazi e i presidi per evitare il contagio nelle aule. Insomma,

determinate questioni che invece andrebbero affrontate caso per caso in quest'Aula, per contemperare nel migliore dei modi il bilanciamento tra interessi differenti.

l'emergenza sanitaria è l'emergenza economica. In effetti è vero: se il Paese non è sano e messo in sicurezza non può riprendere;

non già quando a marzo dello scorso anno ci fu l'emergenza conseguente alla pandemia, ma sulla gestione e sull'organizzazione della fase vaccinale. Avevamo infatti tutto il tempo il tempo necessario e disponibile per poter agire anche in forma legislativa, intervenendo sull'articolo 32 della Costituzione. Il Parlamento, il legislatore non l'ha fatto. Non l'abbiamo fatto e oggi siamo sostanzialmente all'interno di un atto amministrativo che ha una debole copertura normativa nella legge di stabilità. Stiamo discutendo, sostanzialmente, di un piano vaccinale

Vengo al punto. La questione è abbastanza evidente: sappiamo che esistono delle priorità, come la vaccinazione degli ultraottantenni contestualmente alla vaccinazione di questi, i piani vaccinali stabiliscono che si possa procedere con la somministrazione del vaccino AstraZeneca

Quali sono i servizi essenziali, come facciamo a stabilire quali sono, a quali leggi di riferimento ci rifacciamo? Sono servizi essenziali i servizi che sono delineati nell'ambito, ad esempio, della legge che regola lo sciopero nei servizi essenziali? quali categorie sono comprese e quali ne sono escluse? Assistiamo ad un paradosso per cui oggi, sempre a macchia di leopardo, in questa nostra Italia, in alcune Regioni vengono vaccinati i magistrati di un distretto e non gli avvocati, che pure partecipano alle stesse udienze, in altre Regioni questo non accade, perché ancora evidentemente non è stato raggiunto un accordo diretto tra la Regione e le singole categorie. Vogliamo parlare di quello che scrive oggi un importante quotidiano

personale in *smart working*, non sanitario, ma amministrativo, che lavora all'interno dei servizi sanitari. *(Applausi)*. Su queste cose chiediamo che il Governo ci metta la testa e anche un po' di ordine.

a mio avviso più rilevanti. Il provvedimento in esame (esauriti i titoli di coda del DPCM *system*, si torni al più presto ai decreti-legge) è l'occasione per riflettere sul cambio di rotta necessario che saprà dimostrare il nuovo Esecutivo, dando prova di avere a cuore la salute e il benessere degli italiani come bene primario e solidale. Ma altrettanto fondamentale è evitare di sperperare risorse; non c'è diritto alla salute senza il dovere della prevenzione e della sostenibilità. È da troppo tempo che, fin qui inascoltati, rimarchiamo che c'è poca attenzione alla prevenzione. Ma, siccome prevenzione non fa rima con fatturazione, si è continuato fin qui a prevedere capitoli di spesa in capo al commissario straordinario non supportati da *benchmark* che ne attestino la congruenza, disattendendo una strategia di efficace contrasto alla diffusione del virus, con un piano nazionale di contenimento in sicurezza delle sue varianti e di monitoraggio delle loro interazioni con il sistema immunitario e i farmaci, attraverso l'appropriata messa a contratto di tutti i fornitori, non solo di vaccini e farmaci, ma per tutti i tipi di beni e servizi. vero infatti che la cura dimagrante imposta al Servizio sanitario nazionale dal 2010 in poi è criticabile, altrettanto vero è che adesso il rischio è il suo contrario, senza ereditare un sistema tecnologicamente "upgradato", che consenta di dare di più spendendo di meno, nello specifico della pandemia senza nemmeno un sistema nazionale strutturato di sorveglianza attiva e genomica e di governo della mutabilità del virus, a garanzia dell'immunizzazione di massa. Siccome siamo nel pieno di una campagna vaccinale azzoppata, questa volta non per mancanza di piano o di vaccinatori, anche se in fase di rafforzamento con i medici di famiglia, ma per mancanza di vaccini, è di tutta evidenza che, se fossero stati fatti contratti molto più stringenti, con clausole ineludibili di consegna non appena ottenuta l'approvazione dell'EMA, che prevedessero una qualche forma di produzione locale in caso di problemi veri o presunti che fossero nei siti produttivi, con penali fortemente disincentivanti l'inadempimento, non staremmo qui a discuterne. Se l'Italia avesse mandato qualcuno stracompetente in contrattualistica internazionale al tavolo delle trattative, non staremmo qui a lamentare la mancanza di vaccini. Non ci resta che confidare nelle maggiori disponibilità delle dosi necessarie per l'ambizioso piano vaccinale. Siamo certi che le competenze che stanno emergendo nel nuovo Governo sapranno farsi valere in ogni sede, compresa la drastica riduzione della decretazione attuativa. La mancanza di una visione complessiva sin qui palesata si è potuta evincere anche sul versante delle altre patologie, che rimarco meritano lo stesso tipo di attenzione del Covid. Continuare a rimandare *sine die* visite specialistiche, *screening* ed esami radiologici e diagnostici non può non comportare un aumento della mortalità e della morbilità (non solo in oncologia), i cui costi sociali ed economici estremamente rilevanti si vedranno nei prossimi anni, insieme al peso degli sprechi che ricadranno sulle spalle delle future generazioni, senza aver preso seriamente in considerazione l'utilizzo di nuove tecnologie già implementabili, con costi di gran lunga inferiori all'ospedalizzazione, che consentono di monitorare da remoto pazienti che allo stadio iniziale, anziché essere ricoverati, possono essere seguiti con cure domiciliari, liberando risorse umane e strumentali da finalizzare al recupero dei programmi di prevenzione secondaria e degli interventi rinviati. Controprova ne è quanto fatto all'ospedale Cotugno di Napoli per monitorare reparti Covid con braccialetti *wireless*, tecnologia assolutamente sistematizzabile a domicilio. Prevenzione, domiciliarizzazione tecnologicamente assistita delle cure, contrasto e contenimento in sicurezza delle varianti che alimentano la pandemia, come noto di esclusiva competenza al livello centrale, il cui puntuale esercizio, in attuazione delle innovative direttrici programmatiche, financo confermate dalla Commissione europea con il piano HERA, consentirà di intervenire a breve anche sul meccanismo di regolazione cromatica, su cui si continua a insistere, tutto incentrato sull'automatismo del cosiddetto RT, mentre è noto da tempo che occorre prendere del pari in considerazione l'incidenza media e l'RDT. Dopo non essere stati ascoltati sin qui nel nostro plurimo grido di dolore per riconoscere ai medici e ai restanti operatori sanitari e socio-sanitari vittime del Covid un ristoro economico, ora certi che l'Esecutivo rifletterà anche su questo argomento, ponendovi rimedio, andando a recuperare il nostro disegno di legge n. supportabile con le risorse derivanti dalla marginalizzazione degli sprechi recentemente emersi. La solidarietà non deve venir meno, soprattutto in momenti come questi, e bisogna saperla dimostrare, non solo a parole. È ora di agire, agire senza indugio nella riqualificazione della spesa.

nella prevenzione e nella lotta al virus e perché introduce un nuovo strumento nella gestione delle vaccinazioni. Si tratta di una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare le attività di utilizzo e distribuzione sul territorio nazionale dei vaccini. Un altro importante lascito del predecessore di Draghi. Non so voi, ma avverto uno strano, ipocrita, vigliacco silenzio nel dibattito politico di questi giorni, da parte sia di alcuni partiti che di alcuni organi di informazione. Fino a poche settimane fa questo provvedimento del Governo Conte sarebbe stato duramente osteggiato da soggetti politici che avrebbero urlato e si sarebbero stracciati le vesti, accusandolo di voler instaurare una dittatura sanitaria o, peggio ancora, di voler affossare il Paese. *(Applausi)*. In questi mesi abbiamo ascoltato gli stessi affermare tutto e il contrario di tutto, pur di ostacolare il lavoro del Governo precedente. È sufficiente ricordare le loro più recenti dichiarazioni per rendersi conto di quanta falsità e ipocrisia si celasse dietro queste contestazioni. Per questi partiti e per i loro *leader* la suddivisione delle Regioni in zone colorate, a seconda del rischio sanitario, rappresentava una follia, generatrice di caos e danni economici immani. Addirittura c'era chi invitava i cittadini a violare queste restrizioni: politici scellerati che hanno fatto propaganda sulla pelle delle persone, pur di cavalcare il loro sentimento di frustrazione e di rabbia. Tutto questo non accadeva mica un anno fa, ma pochissime settimane fa e adesso - *puff*! - tutto scomparso. O meglio sono scomparse solo le polemiche e il caos, non le fasce di rischio colorate, che erano invece, a detta loro, la causa scatenante. Oggi quindi sappiamo con certezza che si trattava solo di propaganda e di attacchi strumentali al Governo. Adesso che le zone colorate non solo sono rimaste, ma addirittura aumentate con l'aggiunta - udite bene - delle cinquanta sfumature di arancione, va tutto bene, benissimo anzi. Mi domando: come starà giustificando questa tripla giravolta la macchina della propaganda di Salvini? Speriamo non con un *post* sulle tagliatelle all'uovo fatte in casa o magari sulla crostata della nonna. Che volete che sia, se tanto a pagare il prezzo più alto sono stati quei cittadini che davano credito alle loro falsità; del resto, sono gli stessi che hanno portato la Lombardia ad essere la Regione con il maggior numero di morti in assoluto. Anche molti governatori delle Regioni del centrodestra pare abbiano archiviato le polemiche. Pochi giorni fa Attilio Fontana, quello del conto milionario in Svizzera nascosto dietro un *trust* alle alle Bahamas, scriveva che il nuovo Governo avrà al suo fianco le Regioni. Ci rendiamo conto? Questi soggetti ora dicono che collaboreranno costruttivamente con il Governo di cui ora fanno parte. Ne siamo felici, ma ci domandiamo: prima che cosa facevano? prima che cosa facevano? Forse lo ostacolavano anche quando lottava per salvare il maggior numero di vite umane? Un ragionamento che non dovrebbe esistere in tempo di pace, figuratevi in tempo di guerra alla pandemia, come il nostro. Ma forse per qualcuno la politica e il consenso vengono prima delle vite umane delle persone. Proprio in questi giorni, Fontana ha istituito decine di zone rosse in singoli Comuni della Lombardia: giustissimo. Peccato che lo abbia fatto dopo aver detto e ripetuto per un anno intero che non poteva farlo; che la che la responsabilità per la mancata chiusura di Alzano Lombardo e Nembro fosse dell'allora presidente Conte; che lui non poteva di fatto istituire zone rosse locali perché non disponeva né dell'Esercito né delle Forze dell'ordine. E ora che il suo partito è entrato al Governo, come d'incanto si è riscoperto in grado di farlo. Mi domando: quante vite avrebbe potuto salvare se, invece di fare becera politica oppositiva a Conte per oltre un anno, avesse semplicemente fatto il proprio dovere di governatore della Lombardia? Per non parlare delle richieste di centralizzazione dei poteri, in tema Covid, giunte in questi giorni proprio da quel centrodestra che nei mesi scorsi ha sempre duramente criticato il Governo chiedendo più poteri per le Regioni. Vi devo ricordare io i dati sbagliati sui positivi Covid inviati per troppe settimane dalla Regione Lombardia al CTS? Neppure su questo mai un'ammissione di colpa o una presa d'atto del disastro fatto. Anche il sistema mediatico, con qualche eccezione ovviamente, ha fatto una giravolta niente male: la stampa di centrodestra si è curiosamente zittita con l'arrivo del nuovo Governo, mentre l'appoggio incondizionato a Draghi ha portato tanti altri giornali a rivalutare molte misure uguali o quasi a quelle introdotte dall'ex presidente del Consiglio Conte. Veniamo all'attualità. È recente la notizia della sostituzione di Arcuri con il generale dell'Esercito Figliuolo come nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid, accolta con un giubilo collettivo che ha unito sia i partiti che fino a ieri erano all'opposizione che tutti i loro organi di informazione. Esattamente come accadde con la caduta di Conte, perché ai contestatori seriali di Conte non importa dei fatti concreti, ma chi occupa le poltrone: attaccano chi toglie voti, potere e denaro (ed io ne so qualcosa). Poco importa se Draghi seguirà la strada di Conte; poco importa se Bianchi porterà avanti il lavoro della Azzolina; poco importa se la medesima proposta di prolungare l'anno scolastico veniva prima derisa ed attaccata se a farla

C'è un altro silenzio tremendo in questo Senato: quello di chi ha provocato una crisi di Governo scellerata nel momento più difficile per il nostro Paese dal dopoguerra ad oggi. E mentre c'era chi lavorava per ricucire questa crisi, lui volava in Arabia Saudita ad elogiare il principe ereditario bin Salman, indicato dall'*intelligence* americana come responsabile della barbara uccisione del giornalista Khashoggi *(Applausi)*, addirittura ad elevare questo regime totalitario a culla del nuovo Rinascimento. In nome di quali interessi lo ha fatto? Di certo non degli interessi degli italiani. Un clamoroso scandalo di cui si parla troppo poco e che riguarda un senatore della Repubblica, stipendiato con i soldi dei cittadini. *(Applausi)*. Un senatore che dovrebbe dimettersi e lasciare la politica per la vergogna che ha fatto calare su tutto il nostro Paese. Mi accingo a concludere, dicendo che le misure contenute nel decreto-legge oggi in discussione non sono l'orgoglio di nessuno; le vorremmo evitare e stiamo lavorando perché ciò avvenga il prima possibile; ma oggi sono misure necessarie, le uniche veramente efficaci per contenere i contagi, almeno fino a quando la campagna vaccinale non avrà fatto calare drasticamente il numero dei malati e alleggerito la pressione sui nostri ospedali. Allo stesso modo, necessari sono i ristori che devono arrivare prima possibile alle famiglie e alle imprese; ristori che ora si chiamano sostegni. Dai, su, è necessario usare la semantica per far credere al proprio elettorato che le cose stiano cambiando. *(Applausi)*. Ristori che sarebbero già sui conti correnti degli italiani se qualcuno non avesse deciso di gettare il nostro Paese nel caos. Concludo, Presidente. Nonostante tutto quello che è accaduto, nonostante il peggio del peggio della politica, andare avanti a lottare è un dovere, proteggere la salute dei cittadini e l'economia rimane l'unica priorità da perseguire; alla propaganda vanno sempre contrapposti l'impegno reale e il senso di responsabilità, gli unici che ci possono fare andare avanti a testa alta. Il virus era, è e rimane...

Dichiaro chiusa la discussione generale. Sospendo la seduta fino alle ore 15 non solo per l'intervento di sanificazione, ma anche per la contemporanea

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15, 2.2, 2.3, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.14, 3.0.15, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,

Mi domando se non era possibile aspettare dieci minuti, in maniera che un senatore della Repubblica potesse esprimere il suo voto. Non eravamo a giocare, non eravamo a fare interviste, ma semplicemente a lavorare.

Chiuso il discorso della Commissione. Ciascuno prenda il suo posto e recuperiamo i voti persi.

parere conforme a quello del relatore, ma per l'emendamento 4.1 il Governo si rimette all'Aula.

alla luce del fatto che sono sopravvenute modificazioni nella popolazione rispetto all'ultimo censimento di dieci anni fa. Il prossimo censimento avverrà fra pochi mesi, ma probabilmente

intervengo per illustrare brevemente lo spirito dell'ordine del giorno G4.101, che nasce dal nostro emendamento 4.2, accolto nello spirito con favore dall'intera Commissione. L'ordine giorno va a sanare e a risolvere la questione aperta da anni per i piccoli Comuni che si trovano in difficoltà in fase di elezioni quando c'è una sola lista depositata il grande impatto degli elettori residenti all'estero fa venir meno il *quorum* per rendere valida l'elezione. Abbiamo trovato una soluzione tecnica che verrà trasposta in un atto normativo nel prossimo futuro questo ordine del giorno ne certifica la soluzione condivisa ampiamente dal Parlamento. È una grossa soddisfazione perché è una battaglia che portiamo avanti da anni.

del Senato. Il nostro emendamento propone semplicemente di cercare di non addossare un peso enorme e a nostro avviso immotivato della filiera della ristorazione, cioè sui *pub,* i bar, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie e quant'altro, che, come lei sa,

Il nostro emendamento 5.0.13 prevede che nelle zone gialle alla filiera della ristorazione possa essere consentito di rimanere aperta fino alle ore 22,

a mezzogiorno e drammaticamente chiusi la sera, perché la gente, non potendoci andare di sera, se ha voglia di andare al ristorante, si affolla nelle ore in cui è consentito e lo stesso vale per le altre attività similari. Col nostro emendamento

Commissione è stato bocciato un emendamento del genere, con il solo voto favorevole di Fratelli d'Italia; ringrazio la Lega (e non altri partiti) che si è almeno astenuta *(Applausi)*. Qui in Aula mi aspetto un passo in più, ma comunque la ringrazio. Tutte le altre forze politiche non hanno neanche affrontato questa questa incomprensibile anomalia: rispetto a tutte le altre attività, l'unica differenza è che la filiera della ristorazione chiude. Nella zona gialla funziona tutto, sono tutti aperti

che la continuità di questo Governo con il precedente possa interrompersi su questo emendamento. Se c'è una novità che viene dal governo Draghi,

punto per punto, con la dovuta attenzione, alle realtà che ci sono nella società italiana.

possibilità che siano rispettate le norme d'igiene, ma invece moltiplica le negatività. Pertanto, signor Presidente, mi auguro che, prima di votare, ciascun parlamentare, che pure ha voluto sommarsi in questa inedita maggioranza, riacquisti la propria libertà di giudizio Signor Presidente, temevo che arrivassimo a questo tipo di richieste. Viviamo tutti un periodo estremamente disgraziato, da tutti i punti di vista, ma arrivare a

agli altri, trovo che sia una discriminazione grave. Purtroppo siamo tutti nella stessa condizione e dobbiamo solo puntare ad uscire da questa crisi il più presto possibile. Queste azioni queste richieste possono solo portare ad una maggiore discriminazione territoriale, sociale ed economica. Sono molto contenta, quindi, del parere contrario del Governo e spero di non sentire più queste

è un tema sensibile per il Gruppo Forza Italia. Voglio ricordare che in tempi non sospetti siamo stati i primi a segnalare l'anomalia per la quale era possibile consentire la ristorazione all'interno delle aziende aziende e non era invece possibile autorizzare la ristorazione all'interno dei ristoranti, pur nel rispetto di tutti i protocolli. Riteniamo, però, che non siano soltanto i ristoratori, i pasticceri e i baristi a soffrire questa crisi e ad avere diritto di lavorare, per non dover scegliere se morire di fame o morire di Covid. *(Applausi)*. Riteniamo che ci sia bisogno di un provvedimento che affronti in maniera strutturale e complessiva la tematica. Possiamo quindi rassicurare il senatore La Russa che il nostro voto di astensione è un impegno a presentare, in un prossimo futuro, un provvedimento organico che tenga conto delle esigenze e delle difficoltà non soltanto dei ristoratori,

ma esattamente un anno fa, per la prima volta nella storia della Repubblica e delle democrazie occidentali, l'Italia - primo Paese rispetto ad altri Paesi europei - adottò un provvedimento di limitazione delle libertà personali, della mobilità, della libera iniziativa economica e anche della socialità delle persone.

Più rallentiamo gli interventi e più tardi finiamo. Fermarsi a chiacchierare lungo le scale non conviene all'Aula, né è segno di rispetto nei confronti dell'oratore.

che questo fosse un atto straordinario ed enorme, un atto fortemente controverso, che fu fortemente criticato da molte forze politiche. Tuttavia non deve sfuggire che nelle settimane successive tutti i Paesi europei, nessuno escluso, seguirono l'esempio dell'Italia, a riprova che la scelta di andare verso le chiusure e verso queste limitazioni era una scelta corretta. corretta. Si sceglieva di non sottovalutare la pericolosità del virus e la velocità con cui poteva diffondersi. A distanza di un anno, il fronte del contrasto alla pandemia è ancora drammaticamente aperto.

In questi giorni le evidenze scientifiche legate alla diffusione del virus e alle nuove varianti delineano un quadro ancora una volta preoccupante,

Tuttavia, nella normalità con cui oggi convertiamo l'ennesimo decreto-legge non c'è nulla di normale e non c'è nulla di scontato. Nell'anno primo dell'epoca del coronavirus le attività turistiche, le attività ricettive e di ristorazione, le palestre, i centri estetici, i negozi di abbigliamento, il mondo dello spettacolo, dell'intrattenimento e della cultura, le attività portuali e le attività aeroportuali con tutte le filiere annesse

Come capirete, si tratta di un valore economico assolutamente insufficiente non solo a garantire un reddito personale o familiare, ma anche a pagare la fiscalità e i costi fissi. Oltre 350.000 piccole e medie imprese (artigiane e commerciali) e professionisti hanno già chiuso i battenti e solo l'ingente utilizzo della cassa integrazione consente oggi di contenere il problema del lavoro e il problema delle professioni. Gli effetti della crisi sono devastanti sul piano della fiscalità generale. Non sfugga a questo Parlamento che l'INPS, nel corso del 2020, ha prodotto un disavanzo di cassa di 20 miliardi di euro, 15,7 dei quali sono dovuti al fatto che abbiamo chiesto all'INPS di intervenire sulle casse integrazioni e sui 600 euro per i professionisti. Inoltre le scuole sono ancora chiuse e i nostri ragazzi procedono con la didattica a distanza; è un danno per l'apprendimento, ma è un danno anche per la socialità delle persone più giovani.

dall'approvazione dello scostamento di 32 miliardi di euro di bilancio (approvato all'unanimità da questo Parlamento e da questa Assemblea), non si sia ancora trovato il tempo e il modo, da parte del Governo, di mettere a punto il provvedimento sui ristori (o sui sostegni, comunque li si voglia chiamare), è sicuramente un cambio di passo; però è un cambio di passo all'indietro. Ci sono 32 miliardi a disposizione da sessanta giorni e il Governo, insediato già da due settimane, non ha dato priorità a questo provvedimento. Non possiamo permetterci di temporeggiare, perché temporeggiare su queste misure vuol dire temporeggiare sulla pelle della gente. Credo, allora, che il tempo e l'esperienza acquisita in questi dodici mesi debbano mettere in condizione il Governo e il Parlamento di agire subito, di aprire, di chiudere, di determinare gli orari e di farlo non più sulla base di ipotesi o di valutazioni di carattere casuale; di agire sui codici Ateco, ma anche sugli orari, sulla base di certezze scientifiche. Cambiare passo vuol dire anche avere il coraggio, come è stato indicato dalla forza politica Fratelli d'Italia, di ripensare, per esempio, le chiusure e le aperture di alcune categorie Ateco e di farlo su base scientifica. Un Paese grande come l'Italia si salva solo se torna a produrre. Non possiamo affidarci né ai ristori, né ai sostegni, né al *recovery fund*. anche se sono tanti soldi, se un Paese non funziona sulla base dell'economia reale, si bruciano subito. Il cambio di passo ci potrà essere solo nella prospettiva che le persone possano tornare presto alla vita normale, a vivere liberamente, a produrre, a fare il proprio lavoro, ad avere la propria socialità e anche ad essere consumatori. Auspichiamo perciò che l'impegno del Governo in sede europea per la campagna vaccinale possa avere il risultato che tutti quanti speriamo e auspichiamo, che possa essere efficace e ottimale, considerata la capacità organizzativa della sanità italiana,

volevo utilizzare un minuto del tempo a mia disposizione per parlare di un fatto increscioso che è avvenuto poco fa e che ha riguardato il senatore Matteo Renzi. Mi all'arrivo di una busta con due bossoli. Io credo che debba essere espressa solidarietà e vicinanza al senatore Matteo Renzi *(Applausi)*, come ha già avuto modo di fare la Presidenza del Senato, come è stato comunicato, con un gesto che è assolutamente da apprezzare. Crediamo che questi fatti siano la spia di qualcosa che non va molto bene. Non è la prima volta che avvengono ma continuano ad accadere. C'è bisogno di riportare -e questo deve essere un invito alla responsabilità rivolto a tutti noi - il confronto politico nel luogo in cui lo stesso deve avvenire. confronto politico anche aspro, su questioni su cui non c'è condivisione, lacerante, ma che mai deve arrivare alla denigrazione, alla campagna d'odio, alla campagna violenta sulla persona. È qualcosa da cui dobbiamo assolutamente proteggere le istituzioni. Questo è un dovere che abbiamo al di là della nostra provenienza, della nostra appartenenza partitica, delle nostre storie personali. personali. La mia vuole essere soprattutto una riflessione che dobbiamo consegnare a noi stessi, provando a invertire la rotta nel confronto politico. Credo che questa legislatura, per le caratteristiche che ha assunto, potrà fornire qualche soluzione in questa direzione. Il provvedimento che oggi ci accingiamo a convertire in legge è un decreto-legge che si inserisce nel solco delle norme che sono state approvate in questo ultimo anno relativamente alle strategie di contenimento dell'emergenza da coronavirus. Ho sentito alcuni interventi in cui si è parlato di una nuova strategia di carattere economico, che assolutamente deve essere messa in campo e che e che il Governo Draghi, come è evidente da ciò che leggiamo e dai provvedimenti che cominciano ad essere strutturati, metterà in campo rapidamente. Oggi a convertire un decreto-legge che continua nel solco dell'attenzione alla messa in campo di strategie e politiche di contenimento del rischio.

di un decreto-legge che, di fatto, prorogava gli effetti dei due principali atti normativi che hanno caratterizzato la strategia di contenimento dell'emergenza, il decreto-legge n. 19 e il decreto-legge n. fino al 30 aprile, di fatto equiparando quei termini alla data della proroga dello stato di emergenza già decisa dal Consiglio dei ministri.

i protocolli per le attività di ristorazione e per le attività economiche e, più in generale, sociali. Con il decreto-legge in esame si prorogano al 30 aprile i termini di scadenza di tutta quella parte normativa che ha caratterizzato l'inizio dell'emergenza nel marzo 2020.

viene data nuova linfa al tema che riguarda la classificazione del rischio sulla base dei famosi colori: una strategia che, anche se discussa in alcuni casi, è diventata in qualche modo patrimonio anche dei cittadini che, attraverso le decisioni assunte riguardo la collocazione della propria Regione in una delle possibili colorazioni, acquisiscono consapevolezza del rischio che, più o meno diffuso, c'è nella propria Regione. Con il provvedimento in esame viene intensificato questo aspetto introducendo dei termini nuovi per la classificazione delle Regioni relativamente alla quantità di contagi ogni 100.000 abitanti, che determinano quei parametri di scenario (scenario uno, due e tre) nel quale le Regioni vengono collocate in base al minore o maggiore rischio di circolazione del virus. Questo è un aspetto che oggettivamente non poteva essere messo in discussione, perché è una base minima di costruzione di tutte le decisioni che il Ministero della salute e, di conseguenza, le Regioni assumono sul proprio territorio relativamente ai divieti di circolazione e alle limitazioni. Secondo me, dovremmo porci qualche dubbio in più su come oggi trattiamo i dati. In questo senso, nel provvedimento che convertiamo in legge, Italia Viva aveva promosso un emendamento per la costruzione di un osservatorio che consentisse l'analisi giornaliera dei dati epidemiologici, perché

di poter avere dei dati che quotidianamente permetterebbero di assumere le azioni conseguenti. Lo ha detto un fisico importante, Battiston,

all'indice RT in pochi giorni di scendere sotto il livello 1. Questo per dire che possiamo cominciare a ragionare anche su delle strategie nuove ascoltando pareri di docenti e figure di riferimento che già operano nel campo dell'analisi dei dati epidemiologici, come appunto nel caso del docente dell'università di Trento Battiston. È un elemento che dobbiamo vedere come un contributo da dare alla discussione; nessuno ha certezze assolute, ma possiamo pensare di lavorare anche in ambiti nuovi e per certi versi inesplorati. Quell'emendamento voleva essere uno stimolo verso questa direzione, e speriamo che il Governo lo possa recuperare

i termini di scadenza per quanto riguarda le politiche delle chiusure, il divieto di spostamento tra Regioni. Infine, vorrei fare un'ultima considerazione importante: si è dibattuto molto

lo scenario che abbiamo di fronte, le decisioni assunte dal Governo Draghi nei primi giorni di vita e il cambiamento avvenuto (nella struttura

tesa a ricostruire un insieme di competenze in grado di affrontare la seconda fase che, dal punto di vista dell'emergenza, è ancora molto grave e preoccupante, ma che deve vederci protagonisti soprattutto nell'ambito della campagna vaccinale, che è la vera via d'uscita che nei prossimi mesi dovrà impegnare il Governo al massimo livello. Crediamo che le nomine che ci sono state nelle ultime settimane consentano di avere una qualche

Collega, la sorta di proletariato della ristorazione che lei ci racconta mi fa venire in mente quella frase di Montanelli

a tutti, e quindi, il proletariato della ristorazione sarebbe comunque garantito a chiunque abbia a disposizione un terrazzino, un marciapiede, una piccolissima struttura, un giardino. Non si preoccupi, collega: anche su questo staremo veramente attenti a non penalizzare nessuno. Stia serena.

lascito del Governo Conte, migliorato, negli intendimenti, integrato, secondo noi semplicemente in linea con la logica di tutti i provvedimenti sin qui adottati, dal primo provvedimento del Governo Draghi che ci troviamo a votare insieme - con ancora una volta sul versante delle costrizioni, sul fronte della limitazione delle libertà di spostamento individuali, di impresa. Agisce solo e unicamente su quel fronte.

Tralasciando tutto ciò, dobbiamo concentrarci sui vaccini. È del tutto evidente che il vaccino resta l'ultimo baluardo per poter uscire dall'incubo. La famosa luce in fondo al tunnel, il famoso sforzo per coprire l'ultimo miglio, in sostanza tutte le baggianate che ci siamo sentiti dire per mesi dal Governo - caro

Vorrei dire meglio tardi che mai. Siamo perfettamente in linea con questa esigenza, tant'è che oggi, signor Presidente, ci chiediamo per quale motivo il nostro Paese si sia contraddistinto per non avere neanche un vaccino in terza fase.

oltre a registrare il *record* dei decessi e dell'abbattimento di PIL, registriamo anche il *record* maledetto di non essere stati capaci a sviluppare un vaccino in terza fase a tredici mesi dall'inizio della pandemia? signor Presidente, *a latere* di questa singolarità, abbiamo la prima industria farmaceutica d'Europa:

Considerato ciò ed essendo l'attuale strumentazione occupata per la produzione vigente, era fin troppo facile dire che dovevamo predisporci per una produzione autonoma nazionale su licenza

coprire le richieste delle Regioni, perché non le autorizziamo in via transitoria ad acquistare sul mercato, da qualunque tipo di fonte di approvvigionamento, i vaccini validati? Perché non lo facciamo?

Una filosofia ispirata alla massima prudenza, alla massima attenzione e alla voglia di non strumentalizzare in senso demagogico la prostrazione, la stanchezza e la paura delle persone. Non Non c'è qualcuno di noi che non sarebbe felice di poter dire ai cittadini che si può abbassare la guardia, che il momento di abbandonare la linea dell'attenzione è arrivato, che si può inaugurare per tutti una stagione di libertà. Tutti vorremmo poterlo dire, ma c'è chi lo dice facendo demagogia e c'è chi evita di dirlo perché pensa che la demagogia sia spaventosamente pericolosa al momento attuale. Questo continua a essere il momento dell'attenzione e della verità e, se dobbiamo dire la verità, dobbiamo dire che la situazione nel nostro Paese, pur non essendo vicina ai livelli di massimo allarme che abbiamo visto alcuni mesi or sono, è ancora molto preoccupante. Non siamo per niente fuori dal tunnel, dobbiamo essere estremamente vigili e mandare messaggi coerenti ai nostri cittadini, accettando i sacrifici che sono necessari per mantenere sotto controllo la pandemia; una pandemia resa più insidiosa dal proliferare di varianti che hanno costretto gli organi pubblici ad assumere un atteggiamento di maggior rigore e che hanno spinto spinto il nostro Governo, nell'ultimo provvedimento annunciato ieri, a effettuare cambiamenti nelle modalità di contrasto per meglio tener conto di questa novità. Penso sia evidente la validità di questo approccio. Credo che sia stato importante ieri dare il segnale che c'è convinzione sul fatto che il DPCM sia lo strumento più adeguato ad affrontare l'emergenza, a patto ovviamente che esso si inserisca all'interno di una cornice che è quella disegnata dai decreti-legge; così è sempre avvenuto da febbraio in poi dell'anno scorso e così dovrà avvenire in futuro. Come Presidente della Commissione affari costituzionali non mi sono mai iscritto al partito di coloro che chiedevano l'assunzione delle restrizioni tramite decreto, per la semplice ragione che soltanto il decreto non è efficace per rispondere tempestivamente alle esigenze di un'emergenza che alle volte richiede reazioni che devono essere messe in campo nel giro di ore. Non nascondiamo le difficoltà che ci sono state per l'approvvigionamento dei vaccini. Tutti sappiamo che per uscire dal tunnel è necessario che ci sia un salto di qualità, quantitativo e qualitativo, negli inoculi. Sappiamo che, per raggiungere l'immunità di gregge, dobbiamo accelerare fortemente il ritmo delle vaccinazioni. Non ci nascondiamo, perché siamo europeisti - e non perché siamo antieuropeisti - che qualcosa non ha funzionato nella strategia che a livello di Commissione europea è stata adottata per l'approvvigionamento dei vaccini. E denunciamo questo fatto perché ci interroghiamo su quali modifiche, anche all'architettura istituzionale dell'Unione, devono essere apportate affinché limiti del genere in futuro non ostacolino l'azione di contenimento della pandemia. Io credo che ci siano tutte le condizioni per poter fare un lavoro efficace nelle prossime settimane, per poter garantire sicurezza ai nostri cittadini e per farlo in condizioni di rispetto reciproco tra le forze politiche e in un clima di unità che, nelle emergenze, non guasta mai. Vorrei segnalare che durante l'esame del provvedimento da parte della 1a Commissione, che ha effettuato il lavoro di analisi e di approfondimento degli emendamenti, sono stati oltre che inseriti i due decreti-legge assunti successivamente,

anche richiamando in servizio, per un periodo predeterminato, cioè per massimo ventuno mesi da oggi, fino al 31 dicembre 2022, i sanitari che sono attualmente in pensione. Credo sia un'azione realistica quella che ispira un emendamento del genere. Siamo in emergenza e l'emergenza richiede appunto misure emergenziali: scusate il bisticcio di parole. Questa misura appartiene a quella categoria e categoria e ci consentirà anche di rafforzare la capacità di intervento anti-pandemico. Mi sembra importante anche l'emendamento che ha ristabilito una parità di trattamento, perché è giusto non fare mai due pesi e due misure, tra la somministrazione di alimenti e bevande all'interno di esercizi privati e la somministrazione di alimenti e bevande all'interno di circoli ricreativi, culturali e sociali. C'era una discriminazione, che ora non c'è più, e penso che tutti dobbiamo esserne contenti. Molto importante

a intervalli regolari, il commissario per l'emergenza invii una relazione alle Camere e si sottoponga a un confronto con i parlamentari. Questa misura, fra l'altro, mi dà l'occasione per richiamare un'iniziativa che la 1a Commissione affari costituzionali, su sollecitazione particolarmente forte del collega senatore Nazario Pagano, ha assunto nei mesi scorsi, per rafforzare l'idea che il Parlamento debba essere centrale nei periodi di emergenza, anche attraverso un organismo apposito, che possa rappresentare un interlocutore valido e incalzante del Governo. Purtroppo, per l'aprirsi della crisi di Governo e per il suo lungo svolgimento, siamo stati costretti a interrompere la trasformazione del

creare le condizioni per un maggiore coinvolgimento del Parlamento sia sempre estremamente giusto. Queste sono le ragioni che fanno ritenere al Partito Democratico importante un voto un voto positivo sul provvedimento in esame, che riguarda anche - come sappiamo - la posticipazione a maggio 2021 del termine entro il quale dovranno tenersi le elezioni, sia quelle suppletive per i seggi da collegio uninominale vacanti per la Camera dei deputati e per il Senato, sia per l'elezione amministrativa nei Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa. In Commissione abbiamo anche preso atto che alcuni alleggerimenti degli adempimenti, disposti durante l'emergenza per le precedenti elezioni regionali, molto probabilmente saranno necessari anche in vista dei prossimi turni elettorali, perché si svolgeranno quando l'emergenza potrà dirsi tutt'altro che conclusa. Per questi motivi ribadisco l'orientamento del Partito Democratico a votare a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 2 del 2021.

Renzi. Mai sottovalutare le minacce: bisogna sempre rispondere e reagire a ogni atto di intimidazione. Ancora una volta, colleghe e colleghi, come è successo più volte in questo anno di pandemia, siamo qui in Assemblea a votare la conversione dell'ennesimo decreto-legge, che approviamo per fronteggiare il Covid-19. a favore, anche perché il decreto-legge n. 2, nella sua articolazione, su cui poi si è innestato il successivo decreto-legge n. 15, è stato approvato dal Governo precedente, che ha operato bene. Il nostro grazie al presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte e ai Ministri tutti, è autentico e non di circostanza. È vero che già dagli interventi che mi hanno preceduto si respira un clima diverso. Nessuno più chiede il MES, mentre il ponte sullo Stretto di Messina si allontana e su quel *recovery fund*, che tanto faceva discutere, abbiamo visto che il presidente Draghi ha confermato, giustamente, che sarà approfondito e completato per quanto riguarda gli obiettivi strategici e le riforme. Anche quegli attacchi ai ministri dell'interno e della salute, Lamorgese e Speranza, sembrano perdere potenza dal momento che la linea sui migranti e sul rigore per fronteggiare l'emergenza sanitaria è condivisa dal presidente Draghi. Anzi, possiamo dire senza essere smentiti che, nell'ultimo Consiglio dei ministri sulle misure anti-Covid, il Governo Draghi ha agito in piena continuità con quello di Giuseppe Conte: l'ennesimo DPCM, questa volta firmato dal professor Draghi, che andrà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, compresa Pasqua, prevede anche zone rosse e stretta sulle scuole. Purtroppo ci attendono settimane difficili; la curva dei contagi sale, i ricoveri ospedalieri anche. Ci avviciniamo rapidamente alle 100.000 vittime; siamo a 98.288 morti dall'inizio della pandemia, a 2.955.434 contagiati. ci troviamo, nell'arco di poche ore, di fronte a Presidenti di Regione che auspicavano l'apertura serale dei ristoranti e che oggi sono invece costretti ad accettare le zone rosse. Il dato che preoccupa ancora di più l'Istituto superiore di sanità è che è diventata prevalente la variante inglese in Italia: la percentuale è al 54 per cento, con più contagi e più ospedalizzazioni. Oggi, colleghe e colleghi, è cambiato il commissario straordinario all'emergenza Covid: Domenico Arcuri è stato sostituito dal generale di Corpo d'armata dell'esercito Figliuolo. Buon lavoro al generale Francesco Paolo Figliuolo e grazie a Domenico Arcuri. Si apre così una fase nuova e spero che nessuno voglia più continuare in polemiche strumentali inutili e dannose per il Paese. Certo, non tutto è filato liscio, ma voglio ricordare che ci siamo trovati di fronte e siamo di fronte ancora oggi alla più grande emergenza che la storia recente ricordi. Ci sono difficoltà nel piano vaccinale, ma il problema era ed è a monte, e cioè il rifornimento dei vaccini - come hanno giustamente detto i colleghi che mi hanno preceduto - con le case farmaceutiche che non hanno mantenuto gli impegni; ritardi dovuti anche ai contratti firmati dall'Europa che evidentemente hanno lasciato ai produttori dei vaccini la possibilità di non pagare pegno. Dunque, buon lavoro generale Figliuolo. Il decreto-legge all'attenzione oggi dell'Aula del Senato ha un obiettivo principale, che coincide ancora una volta con il rafforzamento della politica di prevenzione dalle infezioni da virus attraverso il principio di cautela. Per questo nel testo sono presenti disposizioni che rinnovano il termine per l'applicabilità di misure restrittive; introducono ulteriori misure circa spostamenti, riunioni, svolgimento delle attività economiche. E non posso non esprimere la nostra più grande soddisfazione per l'approvazione in Commissione dell'emendamento proposto dai senatori del Gruppo LeU e dal sottoscritto, che equipara le attività di somministrazione di alimenti e bevande dei circoli ricreativi, culturali e sociali del terzo settore a quelle di bar e ristoranti. Nel decreto-legge si prevede anche l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale - questo sì che è un elemento di novità importante - per agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali e dei dispositivi e il relativo tracciamento. Solo pochi giorni fa, il 20 febbraio, abbiamo celebrato la prima Giornata nazionale per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da coronavirus. Oggi la situazione internazionale continua a essere preoccupante: i numeri che ci arrivano dalla Francia e dalla Germania non tranquillizzano;

dall'inizio della pandemia, il più alto dato al mondo, più delle vittime di due guerre mondiali e del Vietnam. Come accade nel resto d'Europa, siamo di fronte a numeri da terza ondata. Si continui, quindi, con equilibrio e moderazione come ha fatto il Governo Conte - a gestire le restrizioni imposte dalla pandemia, avendo sempre come obiettivo fondamentale la tutela della salute degli italiani, perché senza quella non può partire nemmeno l'economia. Nelle comunicazioni rese alle Camere il presidente Draghi ha molto insistito sulla priorità assoluta del piano di vaccinazione perché possa essere il più rapido ed efficiente possibile anche per l'approvvigionamento. Ho condiviso, perciò, pienamente le indicazioni che ha dato per accelerare e produrne anche nel territorio nazionale impostando una nuova strategia per reperire un numero di dosi adeguato. A marzo è già previsto l'arrivo di massicce dosi dopo i 4 milioni di febbraio e i 2 di gennaio. Nel secondo semestre sono attese ulteriori forniture. In questo senso è anche importante l'accordo appena sottoscritto tra il Ministero della salute e tutti i medici di medicina generale per somministrare il vaccino Covid, consentendo al nostro Paese, quando aumenteranno le dosi a disposizione, di rendere più forte la nostra campagna di vaccinazione. Sui vaccini occorre fare tutto il possibile per garantire la tutela del diritto alla salute. Bisogna battersi per la questione dei brevetti,

L'epidemia ha cambiato il mondo; ha già avuto ripercussioni drammatiche nel nostro Paese, al di là dell'aspetto sanitario. In questi mesi, con il Governo Conte, si è lavorato per evitare che l'emergenza sanitaria si trasformasse in emergenza sociale, ma questa c'è. Proprio l'Istat l'altro giorno ha confermato che, nel 2020, il prodotto interno lordo è calato del 8,9 il Mezzogiorno appare sempre di più l'area più debole sul piano socio-economico e le previsioni e il rischio di un aumento della cassa integrazione alla fine del blocco di licenziamenti sono più che mai evidenti. Vorrei sottolineare che il motto «Prima il Nord» ha bloccato la crescita del nostro Paese prima della pandemia. Oggi più che mai bisogna ridurre il divario tra Nord e Sud, altrimenti non se ne uscirà. non riparte il Sud, l'Italia non riparte. Signor Presidente, Governo, colleghe e colleghi, siamo in un momento difficile e a noi tocca continuare ad assumere scelte di responsabilità e rigore a tutela della collettività. Concludo annunciando il voto favorevole al decreto-legge in esame dei senatori di LeU e della maggioranza del Gruppo Misto. Prima le persone!

Grazie, segno di evidente intimidazione, ma anche di spregio a questa altissima istituzione credo sia un fatto gravissimo che vada assolutamente stigmatizzato. Aggiungo che quando accadono queste cose bisogna anche domandarsi il perché, quindi è ovvio che dei mandanti morali evidentemente ci sono e noi, che siamo il presidio della democrazia di questo Paese, dobbiamo ricordarcelo sempre e questa è la ragione per la quale oggi lo rammento. Detto ciò, vorrei adesso concentrarmi, com'è giusto che sia, sulla dichiarazione di voto di Forza Italia su questo ennesimo decreto-legge che allunga i tempi

per motivi sanitari, visti i tanti morti. Vorrei fare un inciso su quanto detto dal collega Ruotolo: è vero che in America ci sono stati tanti morti (500.000), ma anche in Italia, presidente Calderoli, abbiamo avuto oltre 98.000 deceduti; 60 milioni di abitanti, in pratica abbiamo una percentuale equivalente a quella degli Stati Uniti d'America, se non addirittura superiore. Se pensiamo che abbiamo avuto 200.000 morti o poco più durante la Seconda guerra mondiale, questo dato fa capire l'impatto terribile

un provvedimento non nasce e si conclude all'interno dell'attuale maggioranza, Forza Italia, almeno in questo, ne prenda le distanze in termini di voto di astensione. Ciò detto, il decreto-legge tratta della zonizzazione del nostro Paese nei vari colori. Non siamo contrari, come abbiamo sempre dichiarato; non ha più senso limitare gli spostamenti, evidenziare certe restrizioni dei nostri concittadini in modo equivalente o comunque identico in tutto il Paese: è giusto intervenire dove esistono e nascono focolai, a maggior ragione a causa di queste terribili varianti, come quella inglese. Per esempio, nel mio territorio di residenza, a Pescara e a Chieti, già da dieci giorni

Fratelli d'Italia, ieri è stato costretto a collocare in zona rossa l'intera provincia di Ancona e non lo ha fatto perché si diverte a realizzare restrizioni, ma perché purtroppo il contagio è cresciuto enormemente anche in quel territorio e non lo possiamo dimenticare, perché ce le dobbiamo dire queste cose.

molto alta, bisogna evitare che vi siano assembramenti. Non possiamo dimenticare le immagini soltanto di pochi giorni fa, in cui a Milano nella zona dei Navigli la gente è impazzita e ha organizzato feste e fatto musica e le persone addirittura si abbracciate le une con le altre. Se abbiamo concittadini che vanno seguiti passo passo, noi, che abbiamo la responsabilità di questi provvedimenti, dobbiamo farlo. Finché non si abbassano la tensione dei

pressante per la società italiana, che è quello dell'emergenza sanitaria, era assolutamente necessario. Il senatore Aimi ha detto in modo abile e corretto, ma soprattutto ricco di elementi

solo utile, ma assolutamente efficace per uscire da questa situazione. Non esiste altra soluzione che quella di vaccinare tutti i nostri concittadini.

proporrà già al Consiglio dei ministri la prossima settimana. L'aspetto legato alla questione dei

che appartengono a questa formazione politica. Noi ci siamo e daremo il nostro contributo. Come sempre, siamo dalla parte degli italiani. membri del Governo, colleghi senatori, anche il Gruppo Lega esprime solidarietà al collega senatore Renzi per il vile atto intimidatorio che ha subito. È già stata emessa una nota congiunta dei nostri capigruppo

Mettiamo subito in chiaro di cosa stiamo trattando e cosa andremo a votare. Al nostro esame c'è la conversione di uno degli ultimi decreti-legge del Governo Conte, l'ultimo tassello di una gestione farraginosa e caotica dell'emergenza Covid. Chiudiamo questa partita e poi voltiamo pagina. La Lega ora c'è e mette a disposizione del Governo Draghi il suo pragmatismo, le sue idee e le sue proposte. Con responsabilità ci mettiamo al servizio del Paese, per riuscire dove Conte e la sua corte dei miracoli hanno fallito. Serve un cambio di passo: innanzitutto è necessario rivedere la tempistica per l'adozione dei provvedimenti, come chiedono anche le Regioni. Serve che imprese e cittadini vengano a conoscere con congruo anticipo se e quando dovranno riorganizzare le loro attività. Basta con la "annuncite" alla Casalino, quella del venerdì sera per la domenica mattina. Per stabilire con maggiore limpidità i criteri per definire le zone rosse, arancioni e gialle serve ridurre il numero dei parametri e semplificare il sistema di classificazione delle zone. Una norma, anche se sgradita, è più facilmente sopportata dalle persone se è chiara e trasparente la *ratio* che l'ha generata. Vogliamo uno Stato amico al fianco dei cittadini, un padre che si prende cura dei figli e non uno Stato padrone che detta ordini incomprensibili. Tra ritorno alla normalità, ripresa delle attività economiche e fondamentale tutela sanitaria, il punto d'equilibrio dovrà essere il buon senso; solo questo dovrà essere il nostro faro. A un anno di distanza dall'istituzione dello Stato d'emergenza, deve ormai esserci la consapevolezza di quali regole e norme funzionino e quali meno, quali siano effettivamente efficaci e quali siano inutili per il contenimento della pandemia, quali abbia senso mantenere e quali vadano cambiate o abolite, perché sono unicamente vessatorie e non producono risultati concreti. A titolo d'esempio, porto alla vostra attenzione il divieto di spostamento tra Regioni gialle o bianche, cioè tra territori aventi lo stesso tasso di rischio. È difficile spiegare ai cittadini che abbiano una qualche minima nozione di geografia perché da Rimini si possa raggiungere Piacenza e non Pesaro, perché da Foggia si possa andare fino a Otranto e non in Molise perché da Bolzano non si possa andare a Trento (distante 60 chilometri), quando da Belluno si può andare a Chioggia (dalle Dolomiti al mare) o da Sondrio si può viaggiare per ore per raggiungere Pavia. Non ci si può spostare dall'Abruzzo al Molise, anche se assieme sono pressoché la metà della dimensione di molte altre Regioni in cui la circolazione è internamente possibile. Tutto ciò è incomprensibile ai più e non fa altro che minare l'autorevolezza e la credibilità dell'insieme delle regole. forse chiara (altra regola difficilmente accettata, perché non spiegata) la logica che obbliga i genitori a non portare con sé per una visita ai parenti, assieme a quelli più piccoli, anche i figli di quindici I *teenager* sono forse la categoria più portatrice di contagi e quindi devono essere lasciati a casa da soli? Se ciò fosse vero, come si concilia questa scelta con quelle relative alla scuola e con le altre situazioni che vedono i giovani protagonisti? Se non c'è una logica, si cambi la norma; se la logica invece c'è, allora la si spieghi bene, se si vuole che venga compresa, accettata e attuata. Vedete, colleghi, al momento la realtà al di fuori di questi palazzi è ben diversa da quella teorizzata dai DPCM. Le famiglie si spostano lo stesso, magari con due automobili, ben sapendo che poi, una volta giunti all'interno delle abitazioni, i controlli saranno pressoché impossibili. Chiediamo più contatto con il Paese reale e meno astrattismi dettati da grigi burocrati. Veniamo a un altro tema trattato dal decreto Conte del 14 gennaio: la piattaforma per la gestione vaccinale prevista dall'articolo 3. Si istituisce uno strumento per monitorare il tracciamento delle dosi di vaccino e degli altri dispositivi e materiali utili. Ci si è preoccupati di come distribuire le dosi, ma il problema era che le dosi non c'erano o, quantomeno, non ce ne sono state in numero sufficiente rispetto ai numeri promessi. Le Regioni si sono attrezzate ed erano pronte a vaccinare in tempi rapidi un elevato numero di cittadini, ma non hanno ricevuto le fiale dal commissario straordinario Arcuri. Bene hanno fatto, quindi, il presidente Draghi a sollecitare la comunità europea e il ministro Giorgetti ad aprire un tavolo con le aziende farmaceutiche nazionali per attivare la produzione nel nostro Paese, per arrivare a un vero sovranismo vaccinale. Bisogna agire e intervenire al più presto, perché è evidente che qualcosa non ha funzionato nella sequenza Big pharma-comunità europea-commissario, magari perché qualcuno era troppo distratto a progettare le "primule". Presidente, dovrei leggere ancora un'intera pagina dedicata ad Arcuri, all'*app* Immuni, ai banchi a rotelle, agli appalti per le mascherine, ma credo che a questo punto, anche prendendo spunto dall'azione del presidente Draghi, si possa soprassedere e stralciare definitivamente tutto tutto quanto riguarda il commissario Arcuri. *(Applausi)*. Ci poniamo, però, un altro interrogativo. Vale la pena creare una nuova piattaforma, quando esistono già i servizi informativi regionali ed è istituita un'Anagrafe nazionale dei vaccini? Non avrebbe più senso potenziare e investire in quelle già esistenti? Dobbiamo infatti considerare che, stante il fatto che è plausibile che i vaccini garantiscano una copertura annuale, con questi anti Covid-19 dovremo convivere per anni. Non sarebbe meglio sin da ora inserire la gestione dei dati nel canale ordinario del sistema sanitario nazionale? Sono interrogativi su cui andrebbe fatta una riflessione. Attenzione e preoccupazione è infine stata espressa dal nostro Gruppo su quanto previsto dall'articolo 5. Il continuo rinvio del termine per il rinnovo agli stranieri dei permessi di soggiorno scaduti comporterà, una volta terminato lo stato d'emergenza, la permanenza sul suolo nazionale di almeno un milione di persone potenzialmente non aventi titolo (al momento abbiamo già superato la soglia delle 700.000), le cui domande di rinnovo verranno esaminate e smaltite in un lungo lasso di tempo. Chiediamo sin d'ora che vi sia quantomeno la previsione di trattare in via prioritaria permessi scaduti entro i primi sei mesi del 2020, per evitare asincronia nel sistema e sperequazioni che favoriscano coloro a cui da più tempo sarebbe scaduto il permesso di soggiorno. Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, sottolineando quanto sia fondamentale che d'ora in poi si abbandoni la logica del doppio binario. Infatti, finora, a un decreto-legge sulle regole ne corrispondeva uno successivo sui ristori, emanato giorni dopo, spesso con effetti ritardati di ulteriori sessanta giorni, connessi alla conversione parlamentare. Ciò lasciava nello sconforto per giorni o settimane chi si trovava dall'oggi al domani a veder venir meno l'unica forma per garantire la sussistenza a sé e alla propria famiglia. Se dovessero in futuro essere previste nuove chiusure, queste dovranno essere abbinate in modo contestuale alle conseguenti misure economiche

alla riapertura progressiva delle attività ora chiuse (ristoranti, teatri, palestre); lo si faccia istituendo, se necessario, nuovi protocolli, anche più rigidi, ma si dia la possibilità a chi vive solo del proprio lavoro di riacquisire la propria dignità. Si può fare con poche regole certe, serie e fatte applicare veramente e severamente: chi le rispetta, resta aperto; chi sgarra, paga e viene chiuso. Signor Presidente, considerate le premesse non condivisibili su cui è nato il provvedimento in esame, risalente al precedente Governo giallo-rosso, che ci hanno portato qualche settimana fa a votare a favore della questione pregiudiziale, ma confidando che d'ora in poi verranno recepite le nostre richieste, cosa di cui abbiamo già avuto dimostrazione con l'approvazione in Commissione di alcuni nostri emendamenti e ordini del giorno, annuncio che il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione

sono particolarmente lieta che mi possa ascoltare la neo Sottosegretaria alla digitalizzazione, perché spero che possano interessare le cose che sto per dire. Il provvedimento oggi in discussione contiene alcune disposizioni urgenti che si applicano al periodo attuale di emergenza epidemiologica e allo svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. Il MoVimento 5 Stelle ritiene fondamentali tali misure e per questo dichiaro subito il voto favorevole del nostro Gruppo. A causa del perdurare della pandemia con le sue varianti, vengono prorogate le misure restrittive che già conosciamo, il cui termine viene spostato dal 31 gennaio al 30 aprile. Dal 20 febbraio, infatti, ha ricominciato a salire in queste due settimane sono aumentati di circa 50.000, equivalenti a circa il 12 per cento in più. Come vediamo e leggiamo tutti i giorni, la situazione è ancora molto seria e non ci possiamo permettere di deragliare dal percorso che abbiamo tracciato in questi ultimi mesi. Si continua quindi a chiudere temporaneamente attività economiche; si chiede di evitare gli assembramenti; si limitano libertà individuali e spostamenti. Purtroppo, si chiudono anche le scuole, con grave danno ai ragazzi e ai giovani per la loro formazione e il loro futuro, ma sono sacrifici ancora necessari. C'è però una rilevante novità che dà qualche speranza, ossia l'introduzione della cosiddetta zona bianca. La situazione odierna non consente neppure lo svolgimento in sicurezza delle elezioni suppletive e amministrative, che per questo sono prorogate da specifiche norme.

e degli altri materiali di supporto alla somministrazione e relativo tracciamento. La finalità enunciata in testa all'articolo è quella di dare piena e celere trasparenza di attuazione al piano strategico dei vaccini. La piattaforma è del Ministro della salute ed è predisposta e gestita dal commissario straordinario, mentre la gestione delle diverse fasi della vaccinazione è affidata alle Regioni e alle Province autonome, che si avvalgono dei propri sistemi informativi vaccinali in qualità di titolari del trattamento. Il punto importante di tale norma prevede, qualora il sistema informativo vaccinale di tali enti non risulti adeguato, che la piattaforma esegua in regime di sussidiarietà le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse. È importante - ed è un deciso passo avanti - che si sia scelto tale regime di sussidiarietà da parte dello Stato. Il livello di prestazione nei confronti dei cittadini viene quindi uniformato, indipendentemente dalla Regione di appartenenza, eliminando i divari territoriali purtroppo ancora esistenti. Da parte del nostro Gruppo sono stati presentati e accolti come impegni dal Governo alcuni suggerimenti veramente necessari perché migliorativi per perseguire il fine della trasparenza espresso nella norma nei confronti dei cittadini, della società civile, della società della ricerca e della scienza. Tramite la condivisione di dati accessibili e in trasparenza, i cittadini potrebbero verificare che le decisioni restrittive vengano prese su basi veramente scientifiche, verificabili, riproducibili e quindi razionalmente accettabili dalla popolazione, anche se costano sacrifici. Solo quando ci sarà una comprensione razionale delle decisioni, sarà possibile avere un'adesione consapevole e sorretta da motivazione condivisa da parte di tutta la popolazione. Pertanto, i nostri interventi prevedono innanzitutto di garantire il pieno coinvolgimento - perché oggi è escluso, ed è un danno - del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione nella fase di attuazione ed implementazione dell'attuale piattaforma nazionale vaccini Covid, oltre che nella creazione di tutte le future piattaforme nazionali, in particolar modo in ambito sanitario. sarebbe molto importante anche nel settore dell'istruzione, tramite la realizzazione di una piattaforma nazionale di Stato per la didattica digitale integrata. Inoltre, bisognerebbe assicurare che tutti i dati riguardanti l'emergenza epidemiologica - con riferimento ai casi, alla situazione delle degenze e all'andamento delle vaccinazioni venissero resi totalmente pubblici, previa anonimizzazione, in formato aperto, disaggregati e continuamente aggiornati, ben documentati, *machine-readable* e facilmente accessibili non solo ai soggetti istituzionali, ma anche alle associazioni della società civile, ai ricercatori, ai *media* e ai cittadini, in modo che essi non abbiano dubbi o perplessità sui metodi di raccolta, elaborazione e presentazione dei dati in frangenti così impattanti per l'intera popolazione. Questo è quanto richiedono oltre 160 associazioni, radunate nella petizione #DatiBeneComune, che ha raccolto circa 50.000 firme. I dati rappresentano un patrimonio per la nostra comunità ed è bene tutelare il loro valore. Questa è l'unica strada per riaffermare l'assoluta competenza degli enti preposti, aprirsi alla totale trasparenza, che è uno dei valori imprescindibili del MoVimento 5 Stelle. Un altro impegno da noi proposto - e fatto proprio dal Governo - consiste nell'inserire nel Piano strategico nazionale, tra le categorie da vaccinare in via prioritaria, anche i medici e i sanitari liberi professionisti, in quanto fortemente esposti al rischio di contrarre l'infezione da SARS-CoV-2, oltre agli informatori scientifici del farmaco, specialisti di prodotto e tecnici che entrano nelle sale operatorie in quanto rientranti nelle categorie prioritarie, poiché assimilabili al personale non sanitario operante a qualsiasi titolo nelle strutture del Servizio sanitario. membri del Governo, colleghe senatrici e senatori, oltre alle misure di questo provvedimento, di fronte a noi abbiamo ancora oggi diverse sfide: la prima riguarda la nuova fase dei ristori (con il nuovo nome di sostegno), che dovranno essere ancora più mirati ed equi, ma soprattutto veloci, perché molti stanno soffrendo a causa di questo ritardo. In particolare, li sollecitiamo a favore di chi davvero ha perso tutto a causa della pandemia e delle nostre imprese che hanno pagato e ancora stanno pagando i gravi danni economici in conseguenza di questa crisi. C'è poi la strategia vaccinale: i vaccini stanno finalmente arrivando; dobbiamo proseguire la campagna vaccinale, che è l'arma più potente per sconfiggere il virus, aumentando sempre più l'efficienza di somministrazione verso i cittadini. La transizione digitale richiede invece di mettere all'opera competenze specifiche di professionisti ben formati e aggiornati rispetto allo stato dell'arte, mentre, purtroppo, troppe volte, nei servizi informatici della pubblica amministrazione assistiamo a superficialità, imperizia e obsolescenza proprio nei passaggi fondamentali necessari a compiere la transizione digitale. Lo denunceremo sempre, finché non vedremo un cambiamento di passo. Infine, c'è il *recovery plan*. Nelle varie Commissioni siamo impegnati in audizioni con tutti i soggetti interessati, in modo da mettere in campo un progetto serio, che ci permetta nei prossimi anni di raggiungere un livello di crescita, di investimenti e di aumento nella produttività che ci possa far superare questa drammatica crisi. In conclusione, colleghe e colleghi, tutto ciò che oggi qui approviamo e abbiamo approvato negli scorsi mesi ce lo chiedono i cittadini, la società civile civile e i nostri bambini e giovani, a cui dobbiamo garantire il futuro: un Paese più innovatore, più scientificamente e meglio organizzato, in cui le giovani generazioni non siano più invischiate nelle pastoie dell'inefficienza, ma possano gioire e fruire di servizi efficienti che li mettano nelle condizioni di uguaglianza a livello europeo e internazionale.

Signor Presidente, come ampiamente previsto, l'auspicato cambio di passo che avrebbe giustificato la fine del Governo Conte-*bis* non si è verificato, smascherando una trama ordita da più attori in funzione di logiche meramente spartitorie. Chi si aspettava i miracoli di un Governo illuminato oggi ha davanti agli occhi solo la brutta copia della gestione precedente. Fa specie, soprattutto, la mancanza totale di riguardo verso la scuola: si sceglie infatti di ripristinare la libertà di asporto anche per le zone rosse dopo le ore 18, il che favorirà assembramenti e quindi diffusioni di contagio tra quegli stessi giovani che si lasceranno poi in didattica a distanza. Sul fronte della scuola, tra l'impegno e il disimpegno, il Governo ha scelto di fare Ponzio Pilato. La scuola, per l'ennesima volta, viene posposta alle attività economiche. In zona rossa, infatti, tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse e ancora non sono pronte le misure dispensative per i genitori che lavorano e compensative per i *gap* di apprendimento degli studenti, salvo poi annunciare il mantenimento delle attività didattiche fino al 30 giugno. Mi viene da chiedere: a distanza o in presenza? È un'operazione sepolcro imbiancato. Tanti docenti fuori sede, inoltre, sono stati tagliati fuori dalle vaccinazioni, perché non rientrano nel piano vaccinale delle Regioni in cui risiedono e nemmeno di quelle in cui lavorano. In altre Regioni, ancora, non è possibile nemmeno prenotarsi per i docenti che operano già in sede sulla piattaforma appositamente nessuno ancora ha posto rimedio. Troppo ampia libertà di gestione delle scuole si lascia, inoltre, ai Presidenti di Regione, già totalmente fuori controllo con la copertura dello Stato, mentre si continua a non chiedere loro conto di quanto abbiano fatto o faranno per garantire l'apertura in sicurezza. È davvero inaccettabile che lo Stato ammetta che l'unica soluzione possibile per le scuole sia quella di chiudere senza che gli enti locali debbano dimostrare alcun tipo di impegno a tenerle aperte. È passato un anno ormai e tanti decreti si susseguono, ma ancora si naviga a vista: cambiano i Governi ed è cambiato chi ieri gridava contro Conte e oggi vota a favore di misure analoghe decisamente peggiorative rispetto a quanto si è fatto in precedenza, mentre quello che doveva essere il quinto decreto ristori è ancora nell'incubatore di Draghi. Per tutte queste ragioni, dichiaro il voto contrario della componente del

della Brexit, annunciava sciagure per i britannici stanno venendo alla luce. Il testardo Boris Johnson, invece, sta avendo ragione. Perché? Per esempio, perché la Gran Bretagna mai si sarebbe sognata di spendere soldi per una miriade di banchi a rotelle, le cui forniture nemmeno sono servite per dare un po' di ossigeno alle aziende del settore del mobile. Mai si sarebbe sognata di far arrivare nelle scuole pacchi e pacchi di mascherine griffate dalla Presidenza del Consiglio e realizzate da un gruppo che fabbrica automobili. Ma, soprattutto, Boris Johnson ha vinto la scommessa sui vaccini, garantendo protezione senza obbligatorietà a tutti coloro che ne avessero fatto richiesta, senza "primule" osannate dalla stampa solo perché disegnate dall'architetto Boeri. Sono stati seri, i britannici. parola oscura a chi ha difeso a oltranza Arcuri, concedendo poteri che non ha nemmeno la regina Elisabetta. Sentiamo dire che Draghi è il decisionista che aspettavamo, perché ha sostituito Arcuri con il generale Figliuolo. Che Arcuri andasse rimosso lo aveva capito anche mio figlio e non c'è bisogno di Draghi per fare cose ovvie. Draghi avrebbe dovuto dimostrare la discontinuità, cambiando il ministro Speranza, il quale è ancora lì con tutto il suo circoletto di consulenti ed espertoni, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. L'imminente nuova chiusura delle scuole è semplicemente vergognosa. State distruggendo le vite dei bambini e degli adolescenti. Il Governo sta reiterando gli stessi errori. È mai possibile che ancora non abbiamo una seria normativa sulle mascherine? Sento dire che ne dovremmo indossare due. Ma chi garantisce sulla loro efficacia? Nessuno. Infatti, un gran numero di mascherine al test di controllo non protegge come dice di fare. Per andare in moto occorre indossare un casco omologato, per andare in giro e proteggersi dal Covid le mascherine sono omologate a spanne. Queste mascherine non servono a nulla; non venite a dirci che vi interessa la salute dei cittadini, perché nei buchi dei controllori stiamo assistendo a vere e proprie truffe che umiliano i cittadini, gli operatori sanitari e soprattutto la verità.

Grazie,

dalle frasi forti e intense pronunciate da un infermiere napoletano, Flavio, che lavora presso l'Azienda Ospedaliera dei Colli. Quel suo ripetere quasi come una triste litania e un grido sofferto di dolore la parola «avvilente» offre la possibilità di una riflessione maturata sia sulla gravità della situazione pandemica, sia sugli sforzi immani e i sacrifici enormi di tutti gli operatori sanitari, di coloro cioè che vivono in prima linea, ogni giorno, nelle corsie degli ospedali o nelle terapie intensive il dramma del Covid-19, l'impatto violento del virus e i danni irreversibili sui pazienti che è capace di produrre. Al tempo stesso, queste parole danno anche un segnale netto e un messaggio chiaro sullo stato di sofferenza interiore e sulle privazioni fisiche che i medici, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari subiscono sulla loro pelle, toccati nel proprio animo per le tante vite umane perse, per chi si poteva salvare e non ce l'ha fatta e per i numeri dei contagi sempre alti e in continuo e costante aumento in questo momento. Purtroppo quello che fa ancora più rattristare ed avvilire, come denuncia Flavio, è il triste contrasto tra il dolore e la sofferenza delle persone colpite dal virus, il loro sconforto, il loro sguardo impaurito e perso nel vuoto, spesso il loro lasciarsi andare e, dall'altro lato, la noncuranza, gli egoismi e il menefreghismo di alcuni che, incuranti delle direttive e dei corretti comportamenti da attuare e da rispettare, necessari per ridurre la diffusione del virus, continuano imperterriti ad avere atteggiamenti completamente sbagliati, a dir poco irresponsabili, dimenticandosi completamente dello spirito di solidarietà e del senso di responsabilità. Avvilente! È un grido di sofferenza che esce dal profondo dell'animo gridato con forza, ad alta voce, quasi per vincere la stanchezza fisica e lo sconforto interiore, denunciando una certa sensazione di avvilimento e di impotenza di fronte al virus e alle sue varianti, più contagiose e aggressive, ma è soprattutto per denunciare il continuo menefreghismo di tanti, spesso sotto gli occhi di tutti noi e per ricordarci che questa battaglia si potrà, sì, vincere con l'aiuto

Signor Presidente, questa mattina, come è stato ripetutamente detto in quest'Aula, è stata recapitata una busta con dei bossoli al senatore Renzi. Secondo consuetudine si apre ora la giostra delle solidarietà per il grave gesto che vorrebbe essere intimidatorio nei confronti di colui che, a testa alta e con la schiena dritta, ha sempre sostenuto le sue idee senza timore degli insulti, rivolti a lui, troppo spesso alla sua famiglia, - devo dire - anche a molti di noi, come capitato anche ieri. Credo però sia arrivato il momento, dentro e fuori questa Aula, di ragionare almeno una volta sul peso che le parole hanno, soprattutto quelle dette in libertà verso le persone che non hanno contezza della corretta dialettica politica e sono pronte a recepire i messaggi, spesso distanti, rivolti a questo o quell'esponente politico. L'episodio di oggi è solo un gesto che ha recepito la campagna di odio che da troppo tempo viene attuata verso il senatore Renzi da parte di coloro che hanno manifestato l'incapacità di raccogliere la sfida politica che lui aveva lanciato; sfida esclusivamente e squisitamente politica. In questo senso in tanti, anche in questa Aula, e anche oggi, hanno risposto solo con un insulto rivolto a Renzi, purtroppo, come dicevo, alla sua famiglia e anche a molti di noi che, consapevolmente, ma anche convintamente, abbiamo aderito alla sua proposta.

oggi le donne in difficoltà diventano renziane. Questo è un *post* di ieri e in troppi sono rimasti zitti di fronte a queste parole. riflessione politica attenta e comune che ci obblighi a riportare il confronto negli ambiti corretti della dialettica politica, rammentando che oggi in tanti, quasi tutti, abbiamo raccolto l'invito del presidente Mattarella ad essere uniti per portare fuori il nostro Paese dalla crisi nella quale annaspa. inutile continuare a recriminare, ad accusare e strumentalizzare qualsiasi episodio che

all'esito di quanto accaduto oggi, afferma che certamente i terroristi di oggi non sono più quelli di una volta. Un altro dice «tagliamogli la testa». Questo è l'effetto che provocano le parole pesantissime che vengono dette; dette; parole in libertà, pronunciate senza sapere cosa si sta facendo. La storia però va avanti inesorabilmente e noi finalmente, tutti noi, chi lo vuole, possiamo essere i protagonisti di un momento che è sicuramente storico. Matteo Renzi ha superato ben altri momenti e, pur esprimendogli tutta la solidarietà, sappiamo che saprà affrontare anche questo disdicevole episodio. Basta però con l'insulto a tutti i costi, basta con l'istigazione

tutto e tutti. Agiamo nell'interesse del Paese, smettiamola con questo clima d'odio, che davvero è totalmente inutile e può sfociare in episodi ben più gravi. Speriamo sia l'ultima volta!

Signor Presidente, come ben noto, lunedì 22 febbraio è franata una parte della falesia sulla quale è ubicato il cimitero di Camogli. Il crollo ha interessato circa 200 sepolture e 320 salme. Alcune decine di bare sono finite in mare. Alla sciagura si è aggiunto l'orrore dello scempio, da parte dei gabbiani, dei cadaveri caduti in acqua. Purtroppo, a distanza di oltre una settimana, non tutti i corpi o loro parti sono stati recuperati. Vorrei qui sottolineare come l'uomo ha da sempre avuto il culto della sepoltura, ma in un'epoca che, sotto molti aspetti, è proiettata alla cruda materialità, non salvaguardiamo i luoghi dove pulsa la vita o, come nel caso in oggetto, quelli sacri della morte. lettura, condividendo pienamente, di alcuni stralci della lettera che la Società geologica italiana ha inviato al Presidente del Consiglio: «Chiarissimo professore, ci permetta di segnalarle l'evento di Camogli come un campanello di allarme di una situazione non più trascurabile. La nostra incapacità di mettere in sicurezza anche i nostri morti ha messo in luce nel modo più drammatico le problematiche di gestione e manutenzione del nostro territorio (...). In questi anni si è lasciato che il nostro territorio invecchiasse, privo delle cure essenziali e necessarie per la sua conservazione. Il territorio è diventato fragile e purtroppo necessita di interventi profondi, incisivi e sicuramente costosi. La vecchiaia del nostro Paese è il cimitero di Camogli che precipita in mare, con il suo bagaglio di memoria e dolore, ma è anche l'inerzia della politica, di fronte alla necessità di una programmazione efficace e continua della manutenzione del territorio Il segnale di allarme di Camogli ci dice che è tempo di andare oltre le emergenze (...). I costi per la riqualificazione del nostro territorio sono un investimento che dobbiamo alle future generazioni, così che il *recovery plan* possa essere l'occasione per invertire finalmente la dinamica dell'intervento straordinario successivo all'evento calamitoso, evitando che l'incuria sia nuovamente la causa dell'innesco di pericoli, che potrebbero trasformarsi in rischi».